colleghi, ieri l'Assemblea generale dell'ONU, con 104 voti favorevoli, 54 contrari e 29 astenuti, ha approvato la risoluzione per la moratoria universale della pena di morte. *(Generali un evento di straordinario valore per l'affermazione dei diritti umani dopo l'adozione, nel 1948, di quei princìpi contenuti nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo di cui ricorre, nel 2008, il sessantesimo anniversario. L'Italia da anni lavora per raggiungere questo obiettivo. Ora, il traguardo tenacemente perseguito dal nostro Paese è stato raggiunto; è stata premiata l'azione del Governo e del Parlamento. L'Italia fu in prima linea nel 1994 quando, per soli 8 voti, la risoluzione presentata dal nostro Paese venne respinta dall'Assemblea generale. Nel 1999 ci fu un altro tentativo. La decisione di ieri dell'Assemblea generale dell'ONU è anche il successo di un metodo. L'Unione Europea ha avuto un ruolo fondamentale. La determinazione unanime assunta dai Ministri degli esteri dell'Unione e il procedere, lo scorso 14 maggio, alla preparazione di una risoluzione sulla moratoria hanno rappresentato il primo passo per la determinazione, nel contesto internazionale, di un nuovo e più vasto consenso per creare le alleanze necessarie per raggiungere quello che oggi possiamo definire uno storico risultato. È stata rilevante l'instancabile attività delle associazioni che da sempre si battono per l'affermazione dei diritti umani e per l'adozione della moratoria universale sulla pena capitale. Il loro impegno ha rappresentato un contributo fondamentale al raggiungimento di questo traguardo. IlParlamento italiano ha stimolato e sostenuto con i suoi atti l'azione del Governo. È un risultato che premia l'Italia, l'Unione Europea e la comunità internazionale che nella sua sede più autorevole è stata in grado di porre l'uomo al centro della sua azione per proseguire il cammino verso l'abrogazione definitiva della pena di morte e la piena affermazione dei diritti umani nel mondo.

Credo che ciò rappresenti un argomento di interesse anche di quest'Aula, che tanto si è dedicata a quel provvedimento. Non vorrei che il decadimento finisse con un «chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto». Al di là delle ovvie conseguenze politiche, se un decreto fortemente voluto dal neosegretario del Partito Democratico viene, per proposta

Sono sconcertato del fatto che le poche centinaia di persone allontanate potranno entro breve tempo rientrare nel Paese o addirittura arrivare a promuovere nuove partenze. Mi chiedo se qualcuno abbia quantificato il danno erariale che ciò ha determinato. Non so se qualcuno si rende conto di quanto costano due mesi di lavoro delle Camere

inammissibile; quando, però, c'è stato l'intervento del presidente Pera, questa ipotesi non c'è più stata perché tutti sapevamo che l'emendamento era privo di significato. A quel punto, il Governo

Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, ad ogni apertura di seduta qualcuno o qualcuna di noi potrebbe alzarsi e dire: ad ogni apertura di seduta qualcuno o qualcuna di noi potrebbe alzarsi e dire: «Oggi è morto un operaio». Questa mattina è morto il sesto operaio dello stabilimento ThyssenKrupp di Torino; ieri ne sono morti cinque in cinque distinti incidenti.

disattenzione, stanchezza, ma questo non basta. Se ciò continua a succedere, vuol dire che alcune vite valgono socialmente meno del profitto;

hanno preso spunto dagli eventi terribili di Ciudad Juarez in Messico dove un'associazione intitolata «*Nuestras Hijas de Regreso a Casa*» (Le nostre figlie di ritorno a casa) a casa) celebra tristemente la scomparsa e la morte di molte bambine rapite e poi ritrovate uccise, torturate e stuprate. Questo ha lo stesso rilievo della pena di morte. Non si può non investire le Nazioni Unite di una tale questione. Non ci accontentiamo più di spiegazioni, anche ragionevoli ma insoddisfacenti. In Italia abbiamo una buonissima legge contro la violenza sessuale che è stata ottenuta

mondiali devono essere investiti di tale questione: non è possibile considerare democratico un Paese in cui le vite dei lavoratori e delle lavoratrici valgono meno del profitto e dove le vite delle donne valgono meno di quelle degli uomini. *(Applausi dai

Signor Presidente, credo che le sue parole sulla moratoria avrebbero meritato un'attenzione più intensa da parte di quest'Aula. Il fatto che ciò non sia avvenuto mi dispiace molto. Volevo però, oltre a questo, segnalare alla sua attenzione e all'attenzione di tutta l'Assemblea e dei rappresentanti del Governo l'esigenza di intervenire immediatamente con una nuova moratoria che dipende da noi, dal nostro Governo e dalle nostre amministrazioni. Da 48 ore 39 bambini dai 2 ai 16 anni e tre donne incinte,

dormono in due furgoni messi a disposizione da singoli privati. L'Amministrazione comunale dice di non avere nessuna possibilità di intervenire. Io credo che, in queste condizioni, al di là della fine che fa il decreto per il quale tanto ci animiamo, ci sia bisogno di un intervento immediato. Si tratta di 39 bambini *rom* di nazionalità italiana e di tre donne incinte che nel V municipio, ormai da 72 ore, si trovano al freddo. Questa è una condizione di barbarie

al suo ruolo di seconda carica dello Stato perché si eviti un'ulteriore violazione alla legalità costituzionale con una possibile reiterazione del decreto-legge sicurezza. sicurezza. Ho notizia che sarebbe intenzione del ministro Amato reiterare il decreto-legge, non sappiamo come e con quali contenuti, ma con una procedura che sicuramente contrasta o può contrastare con quanto 11 anni fa ha stabilito la Corte costituzionale. Mi rendo conto che si cerca di coprire la vicenda del ritiro del decreto-legge sulle ragioni di efficacia giuridica dello stesso ma il problema è tutto politico e ribadisco che se si fossero rispettate le regole di funzionamento del Senato e le procedure sull'ammissibilità l'irricevibilità degli emendamenti questa vicenda non si sarebbe verificata. Quest'Aula, Presidente, insieme a lei - e me ne dispiaccio - ha una rilevante responsabilità, perché avrebbe dovuto e potuto chiudere la vicenda su questo benedetto richiamo all'articolo 13 del Trattato di dichiarandone l'incomprensibilità, ma anche l'inammissibilità per estraneità alla materia. Riflettiamo su quanto è accaduto, perché le ragioni sono politiche. Lei, Presidente, ha piegato alle ragioni politiche le sue funzioni istituzionali.

su quello che è un vero e proprio scandalo: mi riferisco all'uso improprio dei mezzi della Guardia di finanza. Come è stato pubblicato sui giornali questa mattina, il vice ministro Visco, nel corso delle sue vacanze a Pantelleria un anno fa, ha utilizzato un guardacoste della Guardia di finanza per recarsi in visita a un sito archeologico, quello dell'antico popolo dei Sesioti, e in quell'occasione, accompagnato dalla moglie e dal figlio, ebbe modo di erudirsi sui sesi preistorici, sulle lische di pesce di 4.000 anni fa e su altri reperti archeologici. Com'è noto, anche altri Ministri di questo Governo, come il ministro Pecoraro Scanio per recarsi da Roma a Mercogliano, in provincia di Avellino, utilizzano gli elicotteri della Guardia di finanza.

i vari emolumenti che riceve come ex presidente dell'IRI, come parlamentare, come Presidente del Consiglio, come ex Presidente della Commissione europea

sul decreto sicurezza. È distrattivo nella manovra finanziaria, perché distrae i fondi pubblici per dare fondi a chicchessia in questo o nell'altro ramo del Parlamento;

di seguire l'attuazione dei provvedimenti e anche l'azione di presenza degli ispettori degli enti preposti per avviare una soluzione diversa. diversa. Credo che sia giusto ricordare questi fatti quando avvengono e che sia assolutamente necessario non trascurare l'impegno quotidiano. Questo lo assicuro all'Aula e penso lo assicurino tutti i colleghi che sono impegnati in tale direzione.

che ritengo la Commissione bilancio possa rapidamente valutare, di aumentare i fondi a disposizione della Commissione d'inchiesta sulle cosiddette

seguirla con attenzione - che riguarda lo svolgimento dei nostri lavori. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri pomeriggio, ha approvato il calendario della settimana corrente e della ripresa dei lavori dopo la pausa per le festività di fine anno. Come già stabilito, questa mattina avrà inizio la discussione generale congiunta sui disegni di legge finanziaria e di bilancio. Nel corso della mattinata, salvo eventuali questioni incidentali (anticipo che è stata avanzata una questione incidentale, già presentata alla Presidenza), non saranno effettuate, salvo questa, votazioni. A conclusione della discussione generale, nella giornata odierna, saranno svolte le repliche e le votazioni degli articoli del disegno di legge di bilancio, al quale non sono stati presentati emendamenti. Per tale fase della discussione sono state ripartite 9 ore e 30 minuti; 20 ore sono state ripartite per le fasi successive. Nel corso della settimana sarà posta all'ordine del giorno la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio per reati ministeriali nei confronti di un ex Ministro e di altri soggetti. A tale proposito la Conferenza dei Capigruppo ha dato mandato al Presidente di valutare, in relazione all'andamento dei lavori, quando procedere alle relative votazioni con procedimento elettronico, al fine di favorire la più ampia partecipazione ai voti, in ragione del *quorum* della maggioranza assoluta richiesto per l'approvazione delle conclusioni della Giunta. In ogni caso, i senatori che non abbiano partecipato alle votazioni elettroniche potranno comunicare i propri voti in modo palese ai senatori segretari, che ne terranno nota in appositi verbali, fino all'ora che sarà stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo. A conclusione delle votazioni finali con scrutinio elettronico dei documenti finanziari, riprenderà l'esame del disegno di legge recante il Protocollo su lavoro e previdenza, sulla base dei tempi già organizzati. I lavori della settimana dovrebbero pertanto concludersi entro la seduta antimeridiana di sabato 22 dicembre. Dopo la sospensione per le festività di fine anno le Commissioni potranno convocarsi a partire da martedì 8 gennaio 2008. L'Assemblea tornerà a riunirsi nel pomeriggio di martedì 15 gennaio. Il calendario della ripresa prevede l'esame dei disegni di legge recanti interventi nel settore sanitario e universitario e modifiche alla legge sull'autotrasporto, nonché il disegno di legge, fatto proprio dai Gruppi di opposizione, concernente lo scrutinio elettorale con sistemi informatici. Nel corso della stessa settimana avrà luogo la relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia e il conseguente dibattito, per il quale sono stati ripartiti i tempi tra i Gruppi. In ogni caso la Conferenza dei Capigruppo sarà nuovamente convocata nella giornata di martedì 15 gennaio per l'esame del calendario dei lavori.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi senatori, il bilancio dello Stato, dopo il passaggio alla Camera, torna al Senato per la sua approvazione definitiva. Il lavoro emendativo svolto dalle deputate e dai deputati non ha prodotto, rispetto agli obiettivi prefissati nella manovra, effetti peggiorativi dei saldi di finanza pubblica. È da segnalare che rispetto alla prima lettura le spese finali dello Stato, così come si deduce dalla lettura della terza Nota di variazioni, si sono ridotte di 559 milioni e, soprattutto, il saldo netto da finanziare risulta migliorato di 471 milioni di euro, in termini sia di cassa che di competenza. Il totale generale della spesa dello Stato, come è detto, in diminuzione, è riportato nell'articolo 20 dell'Atto Senato n. 1818-B

dopo il passaggio alla Camera e, per quanto riguarda la cassa, di 752.272.438.043 euro, con eguale cifra in diminuzione. Questa riduzione incide quindi sull'articolo 2, comma 7, del disegno di legge e riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Signore e signori senatori, se avrete la pazienza di confrontare i grafici e le tabelle sinottiche che integrano la documentazione a vostra disposizione, sarete in grado di verificare facilmente le variazioni assolute e percentuali della spesa dello Stato suddivisa per missioni ed apprezzare di conseguenza come è cambiata la composizione della torta del bilancio.

È evidente che le quattro tavole cui mi sto riferendo sono solo uno dei possibili strumenti di sintesi per rendere più facile e snella la lettura del bilancio; esse purtroppo scontano i ritardi di una riforma delle procedure di formazione del bilancio che stenta a decollare. In particolare, la sfasatura tra le spese organizzate per missione e quelle più tradizionali dei Ministero, ricapitolate nelle tabelle allegate alla legge di bilancio, offre lavoro interessante anche ai più abili solutori di problemi enigmistici. Segnalo come caso esemplificativo le spese per la Difesa. A me sembra evidente che la vera percentuale di incidenza di questa missione, certificata oggi al 3,88 per cento del totale delle spese del bilancio, in riduzione dello 0,78 per cento dopo il passaggio alla Camera, vada integrata almeno con i 2.974.491.000 euro che la missione 33 (Fondi da ripartire) destina appunto alla Difesa per utilizzi che la pur copiosa documentazione in nostro possesso non chiarisce con immediata evidenza

come gli scorsi giorni ci ha ricordato ancora una volta il Presidente della Repubblica con il suo richiamo a progredire con maggiore speditezza in quella direzione. Va comunque riconosciuto ai colleghi della Camera di aver introdotto in finanziaria (attuale articolo 3, commi da 67 a 71) strumenti e impegni temporali che dovrebbero migliorare l'analisi e la valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, il monitoraggio della spesa di ogni Ministero da parte del Parlamento e il controllo strategico nella pubblica amministrazione. È continuato quindi un lavoro paziente in favore della semplificazione, la chiarificazione e il controllo delle procedure di formazione del bilancio. In conclusione, signor Presidente, non mi resta che associarmi all'auspicio con il quale il collega onorevole Andrea Ricci, relatore sul bilancio alla Camera, ha chiuso la sua relazione all'Assemblea, che il processo di riforma delle procedure di formazione del bilancio dello Stato, oggi soltanto iniziato, possa proseguire speditamente e che il Governo, nell'ottica di un leale spirito di collaborazione istituzionale e nel pieno rispetto delle potestà e delle prerogative istituzionali riconosciute al Parlamento, confermi il proprio impegno in tale direzione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione bilancio del Senato ha concluso positivamente i suoi lavori in terza lettura della legge finanziaria per il 2008, tornata al Senato nel testo approvato dalla Camera dei deputati con tre voti di fiducia su altrettanti maxiemendamenti presentati dal Governo, dopo la conclusione dell'esame nella competente Commissione. Si tratta di un testo che contiene molte integrazioni, aggiunte e modifiche rispetto a quello licenziato dal Senato in prima lettura il 15 novembre scorso. Dico subito, però, che l'impianto della legge che era uscito dall'esame della nostra Commissione e dell'Aula del Senato, a seguito di un confronto di merito molto approfondito e puntuale, rimane sostanzialmente immutato, con alcune limitate variazioni che non incidono in misura rilevante sulla struttura e sugli effetti finanziari delle norme che abbiamo qui approvato. L'esame condotto dalla Commissione bilancio della Camera, poi rifluito con diverse modifiche nei tre maxiemendamenti che compongono il testo a noi trasmesso, si colloca, quindi, in gran parte in funzione integrativa del testo del Senato, con molte norme aggiunte, diverse anche di un certo impatto sostanziale e finanziario, e limitate modificazioni del testo Senato. Le due letture, pertanto, unitamente all'intervento propositivo conclusivo del Governo, si sommano e si integrano tra loro dentro un unico disegno di politica economica e di bilancio che oggi siamo chiamati a valutare e riesaminare. È utile preliminarmente richiamare e commentare gli effetti finanziari delle modificazioni approvate dalla Camera dei deputati, nei modi che ho sopra indicato. La manovra lorda - pari, com'è noto, alla somma delle maggiori spese e delle minori entrate - registra un incremento, dopo la lettura della Camera, di circa 2,2 miliardi di euro, che sommato all'incremento registrato dopo l'esame in prima lettura del Senato (pari a 1,9 miliardi di euro), porta a circa 15,5 miliardi di euro il suo importo complessivo, con un aumento di circa 4,5 miliardi rispetto all'importo iniziale, che era pari a circa 11 miliardi di euro. È bene sottolineare che tale espansione della manovra lorda è stata più che compensata dalla maggiori risorse reperite nel corso dell'esame parlamentare, al punto da determinare effetti addirittura migliorativi in termini di saldo netto da finanziare, per circa 470 milioni per l'anno 2009 e 270 milioni per l'anno 2010. Infatti, le compensazioni reperite a copertura dei maggiori oneri si sono in larghissima parte concentrate su ulteriori riduzioni di spesa, mantenendo pressoché inalterata la pressione fiscale, a testimonianza che l'intervento correttivo del Parlamento non solo non ha abbassato il profilo di rigore della manovra originaria, ma lo ha perfino rafforzato. Sbaglia pertanto chi sostiene che l'esame della legge finanziaria da parte del Parlamento ha aumentato la spesa. Trattasi di una valutazione non vera. In particolare, con In particolare, con riferimento all'espansione della manovra lorda operata dalla Camera, essa è stata compensata per ben 1,8 miliardi di euro da riduzioni di spese e per solo 400 milioni di euro da aumenti di entrata, connessi a misure riguardanti l'accisa sui tabacchi, la vendita dei servizi infragruppo, l'imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni aziendali. Ad essere finanziati per tali importi sono stati, sul lato delle entrate, detrazioni fiscali a beneficio delle famiglie numerose, riduzioni di aliquota

di 500 milioni di euro. Si sono inoltre stanziate risorse aggiuntive a favore del trasporto pubblico locale (400 milioni di euro), per l'accelerazione degli interventi in materia di viabilità e ferrovie e il finanziamento di nuovi interventi su trasporti e autotrasporto (400 milioni di euro), per nuovi interventi in campo sociale e per la gestione delle calamità

tanto in termini contabilistici quanto sotto il profilo politico, è utile sottolineare, ad esempio, l'effettiva portata dell'operazione effettuata dalla Camera sul trasporto pubblico locale. Infatti, le risorse a tal fine destinate, complessivamente pari a 1,75 miliardi di euro, solo in parte sono riconducibili a poste già esistenti in bilancio mentre per la restante parte derivano dall'aumento della compartecipazione delle Regioni alle accise sul gasolio, nell'ambito di un'operazione finalizzata non solo ad alimentare il nuovo fondo per lo sviluppo del trasporto pubblico locale, ma anche ad accrescere il grado di federalismo fiscale, attraverso lo spostamento verso il territorio

sulle autovetture aziendali, per 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Tale riduzione, giustificata dalle minori richieste di rimborso pervenute rispetto alle stime iniziali, incide esclusivamente sulle regolazioni debitorie previste per gli anni indicati. In tal senso, non libera risorse aggiuntive spendibili nell'ambito della manovra, ma consente tuttavia di risparmiare sulla spesa per interessi, in relazione al minor fabbisogno derivante dalla riduzione di autorizzazione di spesa, per un importo valutato in 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che la manovra destina al Fondo per interventi strutturali di politica economica. posto in Commissione il tema dell'approfondimento nel prossimo futuro dell'esatta quantificazione a consuntivo di tale importante posta di regolazione debitoria che ammonta a 17 miliardi di euro. Quanto alla composizione della manovra, l'esame parlamentare non ha cambiato significativamente l'originaria proporzione tra riduzione netta di entrate e aumento netto di spese, almeno per il 2008 e il 2009, spostandola leggermente a favore dell'aumento di spese solo per il 2010. In particolare, la componente della manovra netta riconducibile ad una riduzione di entrate si mantiene per il 2008 intorno al 40 per cento della manovra complessiva, e per il 2009 al di sopra dell'80 per cento, con un lieve incremento rispetto all'impostazione originaria originaria del provvedimento. Le spese e le entrate dunque, pur essendo significativamente variate nel corso dell'esame parlamentare, si sono compensate prevalentemente al loro interno, senza mutare la la fisionomia della manovra. L'esame parlamentare ha semmai lievemente ridotto l'entità complessiva della manovra netta, con un miglioramento dell'indebitamento netto, rispetto al testo presentato dal Governo alle Camere, I tagli di spesa, in particolare, sono cresciuti significativamente durante l'*iter* parlamentare, passando dai 4,7 miliardi del testo iniziale a 5,7 miliardi dopo l'esame del Senato, per arrivare infine a 7,9 miliardi di euro dopo l'approvazione della Camera, con un differenziale di circa 3,2 miliardi di euro tra il testo del Governo e quello oggi in approvazione. A fronte di ciò, anche le spese sono corrispondentemente cresciute, per un importo che tuttavia si è mantenuto inferiore ai maggiori tagli di spesa, determinando una riduzione lieve, ma non trascurabile - pari a 96 milioni di euro delle maggiori spese tra il testo iniziale del Governo e quello oggi in approvazione. Anche dal lato delle entrate si è registrato un aumento, sia pure di entità molto più contenuta ma esso si è mantenuto minore del miglioramento complessivo del saldo, non avendosi, quindi, aumenti di entrata destinati a finanziare maggiore spesa, almeno per gli anni 2008 e 2009. In definitiva, il consistente aumento della manovra lorda non incide in misura rilevante sui saldi fissati nella nota di aggiornamento al DPEF e nel disegno di legge originario, che anzi risultano migliorati, sia pure in misura lieve. Rimangono, dunque, confermati gli obiettivi fissati per il 2008 e per gli anni successivi nel contesto di un quadro strategico finalizzato a favorire la crescita economica, la stabilità macroeconomica e l'uguaglianza sociale. Il *deficit* risulta fissato al 2,2 per cento del PIL per il 2008, ben al di sotto della soglia che aveva determinato lo sforamento all'origine della procedura comunitaria d'infrazione per *deficit* eccessivo. Il debito pubblico accelera la sua discesa dal 105,1

Si tratta di dati inconfutabili che si collocano dentro un percorso virtuoso di risanamento finanziario, di stabilizzazione ed avvio della riduzione della pressione fiscale, di riqualificazione della spesa pubblica anche mediante la sua incisiva revisione, di sostegno alla crescita e di contrasto

punti di PIL, la gestione del bilancio era stata improntata a criteri di creatività e di indulgenza, a misure temporanee che nel periodo 2002-2005 erano state pari a 64 miliardi di euro. Nel corso del dibattito in Commissione è stato sollevato, tra gli altri, un tema di una certa rilevanza per il futuro, peraltro già segnalato all'inizio della sessione di bilancio da parte del Ministro dell'economia.

che il finanziamento di nuovi obiettivi, di spesa o di riduzione della pressione fiscale va conseguito con ulteriori incisivi interventi sul lato della riduzione e della qualificazione della spesa pubblica. Ciò è tanto più evidente se si considera l'effetto, sotto tale profilo, della norma contenuta al comma 4 dell'articolo 1 (quello, cioè, che destina l'extragettito alla riduzione della pressione fiscale in favore dei lavoratori dipendenti), che nel testo approvato dalla Camera, che autovincola quindi il Governo e il Parlamento a destinare l'eventuale extragettito del 2008 alla riduzione, appunto, delle imposte per i dipendenti, si riferisce non alle eccedenze di gettito rivenienti dalla lotta all'evasione, ma all'extragettito nella sua globalità. Se questa è la via, è evidente che il Governo e il Parlamento dovranno attrezzarsi per tempo. Si dovrà proseguire sulla via intrapresa dal Governo con la *spending review* e le Commissioni bilancio delle Camere potranno e dovranno partecipare per tempo a tale lavoro, come ha proposto e sottolineato il presidente Morando in Commissione. Per svolgere bene tale lavoro, potranno tornare utili, oltre al lavoro già impostato dal Governo, le norme che sono state introdotte alla Camera ai commi 67 e seguenti dell'articolo 3, cui faceva riferimento poc'anzi il senatore Albonetti, che prevedono attività ben precise del Governo e di altri organismi tecnici, quali: programmi di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, la redazione di una relazione sullo stato della spesa e sull'efficacia nell'allocazione delle risorse da sottoporre alle Commissioni parlamentari ed altre attività finalizzate a rafforzare la ristrutturazione del bilancio dello Stato (già avviato quest'anno in via sperimentale) e ad accrescere le capacità complessive di analisi conoscitiva e valutativa del bilancio stesso. Ricordo all'Aula che in particolare quest'anno abbiamo sperimentato quanto sia difficile per le strutture del Governo fornire elementi valutativi sugli effetti finanziari di talune misure. Lo abbiamo verificato allorquando abbiamo posto al Governo il tema degli effetti, ad esempio, delle misure di risparmio sulla gestione degli immobili pubblici, sul tetto alle retribuzioni dei *manager* pubblici, sulla soppressione degli ATO e diverse altre norme di cui andavamo proponendo l'introduzione.

del Garante per la sorveglianza dei prezzi; riforma - come anticipato - del trasporto pubblico locale; Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa; riforma della modalità di determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; misure per la sicurezza con aumenti significativi di fondi; misure per l'ambiente e la protezione civile, per le calamità naturali e i terremoti, per la valorizzazione degli immobili pubblici con un nuovo meccanismo molto interessante affidato all'Agenzia del demanio; nuova disciplina sulla gestione dei residui di bilancio dello Stato; sostegno alla stipula di mutui per privati ed enti locali per il recupero dei centri storici;

(sicuramente positive e virtuose), razionalizzazione e contenimento dei costi della rappresentanza negli enti locali, nelle comunità montane, accanto ad altre misure come la *class action,* le assunzioni nella pubblica amministrazione, l'aumento dei fondi per il 5 per mille, limitatissime modifiche alla stabilizzazione dei precari e al tetto sui *manager* pubblici ed altre ancora contenute analiticamente nella relazione che consegnerò a conclusione del mio intervento. Il testo che esaminiamo in terza lettura può considerarsi nel suo complesso positivo ed idoneo a conseguire gli obiettivi di politica economica e di bilancio che ho richiamato all'inizio. Su un punto ritengo necessaria una riflessione conclusiva: quello delle dimensioni quantitative dell'articolato e della natura delle norme introdotte nella pregressa doppia lettura, tema sottolineato in particolare dalle opposizioni in Commissione. Sulla scorta dell'esperienza dello scorso anno, del lavoro approfondito condotto dalle Commissioni bilancio di Senato e Camera sulle ipotesi di riforma degli strumenti di bilancio, delle innovazioni introdotte dal Governo, anche relativamente alla struttura del bilancio e della legge finanziaria, la sessione di bilancio di quest'anno si era avviata sotto l'auspicio di licenziare un testo più snello e più leggibile. Purtroppo, tale intento è stato conseguito solo in parte, essendo evidente che le dimensioni e la struttura del testo ci hanno anche quest'anno disvelato le difficoltà del Parlamento di contenere gli interventi entro il limite auspicato, all'inizio della sessione di bilancio, anche dalle più alte magistrature dello Stato. Il problema non è evidentemente risolvibile soltanto coltivando le buone intenzioni o esorcizzando la spinta emendativa da sempre proveniente dal Parlamento, anche a causa delle difficoltà di garantire celerità ed efficacia al normale procedimento legislativo in corso d'anno. un intervento riformatore più incisivo le cui linee essenziali sono state scandite con il documento conclusivo approvato dalla Commissione bilancio nella scorsa primavera, all'esito del confronto cui mi sono sopra riferito, che consenta di affrontare più incisivamente anche il tema degli interventi normativi settoriali e territoriali, Credo, comunque, che possiamo rivendicare la qualità del lavoro che sul punto è stato fatto in questo ramo del Parlamento, in gran parte determinato dalle decisioni del Presidente della Commissione in ordine al contenuto proprio della legge finanziaria all'origine vagliato, ai criteri di ammissibilità ed alla fissazione di termini inderogabili anche per il relatore e il Governo per la presentazione degli emendamenti in Commissione e in Aula. Tali decisioni, anticipatrici dell'auspicata riforma, unitamente al senso di responsabilità e alla qualità del confronto espressi sia dalla maggioranza che dall'opposizione, ci devono far ritenere soddisfatti del lavoro che abbiamo svolto e che la Camera - che pure ha positivamente concluso l'esame in Commissione bilancio non ha potuto svolgere appieno sia per ragioni regolamentari che per la diversa condotta politica della maggioranza e dell'opposizione. Pur tuttavia, la doppia lettura quest'anno ha consentito un vaglio parlamentare serio ed approfondito della manovra sia al Senato che alla Camera, dopo anni di blindatura del testo con un unico maxiemendamento del Governo a seguito della mancata conclusione dei lavori nelle Commissioni. Ciò deve da un lato farci apprezzare positivamente il lavoro complessivamente prodotto dal Parlamento e dal Governo, dall'altro può consentirci di concludere che il confronto parlamentare è stato serio ed approfondito. onorevoli colleghi, nella consapevolezza che il testo della legge finanziaria che ci accingiamo a riesaminare costituisce il frutto di una sintesi e di un confronto democratico tra Governo e Parlamento, nella maggioranza e tra questa e l'opposizione, ve ne propongo l'approvazione nel convincimento

e si erano fatti buoni propositi di non peccare più l'anno successivo: si era addirittura parlato di una sorta di convenzione istituzionale tra il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio e i Presidenti dei due rami del Parlamento per asciugare il testo. Ebbene, il risultato è sotto gli occhi di tutti: la finanziaria è partita con 97 articoli, ha subito qualche passaggio parlamentare; ci troviamo adesso con circa 1.200 commi, che rappresentano il secondo *record* storico vanno assolutamente in deroga alla norma di contabilità di Stato, perché recano norme di carattere microsettoriale, localistico che non hanno nulla a che vedere con gli effetti finanziari. Praticamente è diventato un *pot-pourri* di qualsiasi cosa. In sostanza, sembra proprio che non ci sia stato nessun controllo da parte di chi avrebbe dovuto avere la responsabilità politica di controllare la finanziaria. Non si tratta di questioni di norme giuridiche o di norme procedurali, ma si tratta di avere una responsabilità politica che quest'anno è sembrata proprio mancare. Signor Presidente, la manovra finanziaria è diventata talmente scolorita che qualche idea che forse buona poteva esistere alla sua base si è andata completamente perdendo perché affogata in un mare di mancette (non so se elettorali, preelettorali, oppure per tenere insieme una variegata maggioranza) che l'hanno resa una vera e propria accozzaglia. al Senato il Governo si era comportato come un *bancomat*, ricevendo qualunque richiesta di finanziamento, ma se al Senato è stato un *bancomat*, alla Camera dei deputati è stato un vero e proprio cassonetto.

squallido spettacolo che è ben descritto nei versi del sommo poeta quando dice: «Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta...» (sappiamo tutti come prosegue). Questa manovra finanziaria ha mancato completamente di un nocchiero in un periodo difficile.

quando questo andamento non è dimostrato. È vero che nel 2007 ci sono state maggiori entrate, come dimostrano i dati contabili; è vero che sprecare queste maggiori entrate per costituire un tesoretto da spartirsi è una pratica che va bene tra i bucanieri della filibusta, ma non va bene in un Paese civile;

che noi siamo in presenza di un probabile calo dell'incremento del PIL nel prossimo anno. Il Governo e gli organismi internazionali e nazionali hanno

il livello delle entrate e le prospettive economiche. Oltre al tasso di crescita, dobbiamo tener presente anche gli effetti dell'incremento del costo del petrolio (che non sono quantificati in misura credibile nel Documento di programmazione economico-finanziaria) e gli effetti della

quest'anno un incremento di crescita dell'IRPEF e dell'IRES molto notevole. Ma perché? Perché c'è stato un aumento della tassazione nominale delle aliquote dell'IRPEF ci sono state misure cosiddette antielusive sulla tassazione delle imprese che hanno portato a far riconoscere come guadagni ciò che in realtà erano spese di produzione. Da qui sono derivati aumenti molto cospicui. Se guardiamo però all'andamento dell'economia vero e proprio, ossia all'andamento dell'IVA, registriamo un aumento in linea con la crescita dei redditi nominali, quindi in sostanza una stasi, che si riprodurrà l'anno prossimo quando non ci saranno i soldi per coprire le ingenti spese che sono state disposte manovra finanziaria. Tra altro, mi si consenta, quando un Ministro dell'economia va dicendo che quest'anno con la finanziaria si restituisce, mentre l'anno prossimo occorrerà varare una manovra di 10 miliardi di euro, cioè 20.000 miliardi delle vecchie lire, mi domando di che cosa stiamo parlando. Se si deve fare una manovra, la si deve fare adesso che l'economia va un po' meglio, non l'anno prossimo quando andrà peggio. Non ha senso rinviare a domani un'azione di risanamento - ammesso che ve ne sia il bisogno - che si poteva fare oggi in condizioni migliori, perché domani sarà sostanzialmente impossibile farla, a meno che - questo è il retro pensiero - non si pensi che domani toccherà a qualcun altro e si va via «avvelenando i pozzi». Credo che sia esattamente quello che sta succedendo. finanziaria non funziona e se non funziona la copertura e d'altronde tutta la manovra si basa sulle maggiori entrate e anche sul risparmio pubblico

Per fare cosa? Posso capire che si fa un sacrificio oggi per compiere un'azione importante come risanare il Paese, dare sviluppo all'economia, far partire le imprese, assicurare condizioni di vita migliori ai ceti più deboli. No, signor Presidente, si prendono i soldi a fatica guadagnati dai cittadini sottraendoli con un'imposizione fiscale crescente - non dimentichiamo che il peso delle tasse sul PIL è aumentato di due punti percentuali da quando sono al governo le sinistre - per distribuire a pioggia delle spese sostanzialmente inutili, per finanziare, a spese dei contribuenti, una maggioranza che non trova una ragione né politica né morale per stare più insieme.

di varare un intervento a favore delle imprese, certo c'è una diminuzione dell'aliquota nominale dell'IRES, ma controbilanciata da un aumento della base imponibile, quindi, sostanzialmente, le imprese continueranno a pagare lo stesso. Mi chiedo se è così che si possono attrarre investimenti nel nostro Paese, se è così che si può risolvere il problema dello sviluppo, che pesa come un macigno sul futuro. Credo, in realtà, signor Presidente, che questa maggioranza, pur di stare insieme e continuare a governare, abbia abbandonato lo scopo principale che deve contraddistinguere un'azione di governo: quello di guardare al futuro, quello di scrollare di dosso al Paese questa cappa di declino che si è pesantemente posata sulle spalle di tutti noi da quando c'è questa maggioranza.

Il giudizio più benevolo che si possa attribuire alla finanziaria varata da questo Governo è quello di una finanziaria assolutamente inutile. Una finanziaria ideologicamente basata sul motto della redistribuzione o del recupero dell'egualitarismo salariale. Signor Presidente, la redistribuzione potrebbe avere senso a condizione che ci sia lo sviluppo perché non si può redistribuire la povertà, bisogna far crescere la torta per darne fette più grandi a ciascuno. Non si può litigare sulle briciole di una torta che si va rinsecchendo di giorno in giorno. Ma mi domando se l'immobilismo sociale, che corrisponde alla visione rigidamente egualitaria della nostra sinistra, abbia più senso in un mondo aperto. Già avrebbe poco senso in un Paese chiuso, che non si debba confrontare con quello che accade all'estero. Forse avrebbe potuto avere senso all'epoca del medioevo o due secoli fa, ma adesso che viviamo nella competizione globale,

conferire in tal modo maggiori possibilità di sviluppo e di benessere alle generazioni attuali e future? Credo che se guardiamo realmente al futuro dobbiamo consentire una maggiore mobilità sociale, una maggiore competizione all'interno del nostro Paese. D'altronde,signor Presidente, quello che fa questo Governo è sostanzialmente creare un serio problema alle classi più deboli perché una politica di crescita così evidente della spesa pubblica e della tassazione ha effetti inflazionistici. Non a caso nel nostro Paese c'è un tasso di inflazione più alto che nei nostri *partner* europei perché sostanzialmente si spende di più per avere gli stessi servizi, quindi ogni servizio viene a costare di più, il reddito vale sempre meno e l'inflazione è la tassa più pesante che colpisce soprattutto i più deboli. Questo è quello che bisogna evitare di fare ed è invece quello che invece si sta facendo. Abbiamo visto che solo per i servizi pubblici gli italiani spenderanno mediamente 2.500 euro in più all'anno, cioè circa

che la maggioranza fa pagare agli italiani incolpevoli. È questo, signor Presidente, il vero costo della politica e non altro! *(Applausi dal Gruppo FI)*. D'altra parte, le misure di contenimento della spesa sono state edulcorate sbandierati tagli ai costi della politica si sono ridotti a qualche risibile misura rinviata nel futuro. Non è rimasto niente di rigore, ma è rimasta solo una norma di spesa dietro l'altra. Ho sottolineato che il punto a tenere insieme la maggioranza. Si tratta di un insieme di regali inutili che non mostrano altro che l'incapacità della maggioranza e del Governo di tenere i cordoni della spesa. Insieme a tutto ciò vi sono norme vi sono norme veramente preoccupanti. Mi riferisco, ad esempio, al comma 94 dell'articolo 3, laddove in tema di assunzione dei precari - sappiamo quanto la norma sia pericolosa per le finanze pubbliche - è stato introdotto all'ultimo momento nel maxi-emendamento governativo un inciso

sbagliate; al comma 334 dell'articolo 2 si arriva ad istituire un fondo di solidarietà per l'accesso possibile alle risorse idriche. Si comprende quanto questa sia una norma ridicola in sé:

Poi c'è un'altra norma che dimostra l'incapacità di comprendere quello che succede nel nostro Paese. Signora Ministra, lei era in Consiglio dei Ministri, penso, quando il Governo ha chiesto la fiducia su questi emendamenti, avete votato la fiducia. Lei, insieme ai suoi colleghi, ha inserito nella norma di fiducia l'attuale comma 344 dell'articolo 2 che leggo, perché magari può essere sfuggito nell'abbondanza di commi. la Camera ha approvato oltre 300 nuove modifiche, un *record* mai visto, senza il minimo controllo, senza che nessuno si curasse di vedere quali erano le cose buone e le cose indecenti. Il comma 344 è indecente e glielo leggo, signor Presidente: «È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato «un centesimo per il clima» nel quale affluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione volontaria di un centesimo di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l'autotrazione, nonché per ogni 6 kW/h di energia elettrica consumata». che i cittadini italiani vogliano pagare un centesimo volontario per ogni litro di benzina comprata? Lei pensa che un governante che sa in che Paese vive

Sa quanto costa un biglietto del tram? Lo avete mai pagato con i vostri soldi? E andate a chiedere agli italiani di contribuire volontariamente con un centesimo sulla benzina? Ma voi sapete in che Paese vivete? Io credo che non lo sappiate, non meritate di governare un Paese che non conoscete, signor Presidente. Detto questo, concludo con l'ultima chicca dalla finanziaria: in un comma, signor Presidente, si cambia l'IVA relativa alla cessione di asini, cavalli, muli e bardotti vivi per la macellazione. Ovviamente la finanziaria è una legge che regola grandi principi, la macroeconomia e quindi si occupa della cessione di asini, muli, cavalli e bardotti.

Presidente, approvare una legge finanziaria in prossimità di fine anno, evidentemente, a causa del numero di commi di cui è composta, diventa un esercizio complesso che mette in difficoltà la società civile e la burocrazia nella sua applicazione. Abbiamo visto quanto sia difficile comprendere un testo, complesso di per se stesso, se poi anche nella forma, e quindi non solo nella sostanza come è stato illustrato dal relatore di minoranza poco fa,

e la limitazione dell'uso o dell'abuso della apposizione della questione di fiducia. Credo davvero che il primo gennaio, ancora una volta, sarà molto difficile comprendere

di una norma che intende obbligare le Camere alla chiarezza nel processo legislativo, in modo che ci sia affinità

è composto di 387 commi, il secondo di 642 e il terzo di 164. Il totale di questa legge finanziaria è

questo sia davvero un limite che rende incomprensibile. Esiste un problema di processo legislativo, questo è sotto gli occhi di tutti, ma è evidente che esiste anche un problema politico, cioè di coesione della maggioranza. La

le opposizioni, con senso di responsabilità, alla luce dell'attuale situazione e per consentire il rispetto della volontà del Presidente della Repubblica, hanno presentato un numero assai

che in questo caso è anche sostanza - ma nella sostanza in senso stretto, perché sul *welfare* questo ramo del Parlamento non potrà dire nulla. Qualcosa è stato detto e discusso al di fuori. Evidentemente, signori, il processo legislativo non si svolge più all'interno di questa Camera che deve solo ratificare questioni che sono state risolte e discusse al di fuori della stessa. Quindi, ai sensi del Regolamento del Senato, signor Presidente, chiedo ai colleghi che venga approvata la questione pregiudiziale che, a nome della Lega Nord, assieme ad altri colleghi, abbiamo presentato.

ho chiesto di intervenire in questo dibattito per porre al Ministro dell'economia e al Sottosegretario alcuni quesiti su aspetti che hanno ispirato la manovra finanziaria e che meritano, a giudizio di chi parla, un particolare approfondimento. Nell'edizione *on-line* del sito «Fisco oggi», notiziario ufficiale dell'Agenzia delle entrate, ho rinvenuto lo scorso 7 novembre un commento relativo alle modifiche che questa legge finanziaria dispone con riferimento particolare alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa. Questo commento si intitolava «Interessi passivi, una stretta che viene da lontano», ed era firmato Michele Andriola, un giovane funzionario dell'Agenzia delle entrate, che opera presso la direzione centrale Accertamento di Roma-Ufficio soggetti di grandi dimensioni. II commento in questione , come dicevo, si proponeva di spiegare le ragioni di «Politica tributaria (con la "P" maiuscola)», così testualmente scriveva l'autore, quasi con una sottile vena di autoironia, che ispirano la scelta di questo Governo e di questa maggioranza di stabilire forti limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi per le imprese, e l'autore sosteneva la correttezza di tale decisione politica alla luce del fatto che la deducibilità degli interessi passivi fino ad oggi ha permesso alle imprese di mettere in piedi espedienti che consentono loro «di non «di non pagare le tasse, senza fare uso di costi per fatture false o senza battere gli scontrini per ottenere profitti in nero». In sintesi, la tesi sostenuta nell'articolo è che gli imprenditori italiani (la generalità degli imprenditori italiani, evidentemente) sostengono interessi passivi non per necessità, avendo bisogno di finanziare la propria attività, bensì per accurata scelta di malversazione fiscale a danno dello Stato, avendo essi i capitali propri necessari, ma preferendo portarli all'estero per percepire lì interessi attivi e proventi non tassati in Italia, che vanno a pareggiare gli interessi passivi pagati in Italia, ma fiscalmente dedotti con conseguente occultamento del proprio reddito. Il Ministero delle finanze per bocca di questo suo autorevole funzionario sostiene quindi che «il nostro imprenditore si è auto-prestato i soldi grazie all'interposizione di una banca estera» e che, quindi, non resta al Governo altra soluzione che stabilire l'indeducibilità degli interessi nella determinazione dei redditi d'impresa. Chi parla, signor Sottosegretario, è rimasto sbalordito e sconcertato dalle inquietanti tesi di questo funzionario dell'amministrazione finanziaria dello Stato, essendo del tutto evidente il pregiudizio ideologico che traspare dalle sue parole verso chi fa impresa in Italia, piccolo o grande che sia. L'articolo citato consente però una volta tanto di cogliere, con rara trasparenza, le reali motivazioni delle vostre scelte in questa finanziaria: gli interessi passivi devono essere resi indeducibili dal reddito di impresa come regola generale applicabile a tutte le società di capitali (anche le più piccole, già vessate dagli studi di settore, nonostante l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria), perché per il fisco la regola generale di comportamento degli imprenditori italiani è quella di fare impresa indebitandosi, non per necessità di sviluppare il loro progetto, ma per volontà di frodare l'amministrazione finanziaria dello Stato. Sono, queste, conclusioni aberranti, degne di un inquisitore spagnolo o di un gabelliere del secolo quindicesimo, piuttosto che di un soggetto preposto ad assicurare il corretto, sereno ed equo funzionamento del rapporto tra Stato e contribuenti. Mi chiedo e le chiedo, onorevole Sottosegretario: ma dove vivono questi vostri funzionari? Sulla luna? È del tutto evidente che questo vostro solerte funzionario non conosce la realtà delle piccole e medie imprese italiane, quelle, per intenderci, che costituiscono il nerbo del tessuto produttivo nazionale e producono la maggior parte del PIL del nostro Paese, e che ogni giorno, con grandi sacrifici, spesso stringendo la cinghia e rischiando l'osso del collo, fanno ricerca, fanno innovazione, combattono sui mercati internazionali per la loro sopravvivenza. Ho pertanto rivolto immediatamente al Ministro dell'economia un'interrogazione, sottoscritta anche da numerosi altri colleghi, per sapere se l'intero Governo condividesse le argomentazioni di questo Michele Andriola e se risulti che le tesi espresse nel citato documento, peraltro pubblicato su un notiziario telematico ufficiale dell'Agenzia delle entrate, coincidano con l'impostazione e le direttive generali che i vertici dell'Agenzia delle entrate impartiscono ai propri funzionari. Naturalmente, onorevole Sottosegretario, nonostante io l'abbia anche sollecitata in corso di seduta, nessuna risposta è stata data fino ad oggi al mio atto di sindacato ispettivo. Perché, onorevole Sottosegretario, non prova ad esprimere lei il suo parere a riguardo proprio oggi, replicando al mio intervento? O teme il severo giudizio dei contribuenti che ci stanno a ascoltando? Queste sono le risposte che gradiremmo avere come contribuenti, prima che come parlamentari, piuttosto che le solite generiche, fumose e inconcludenti dissertazioni su queste norme che puniranno, senza ragione alcuna, la piccola e media impresa italiana. Pochi giorni dopo l'articolo di Andriola, il dottor Fabrizio Carotti, capo del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia, ha rilasciato ad un importante quotidiano economico nazionale un'intervista, nella quale anch'egli spiegava e difendeva le scelte concernenti il nuovo assetto della deducibilità degli interessi passivi dalla base imponibile IRES, delineato in questa legge finanziaria. Ho provato ad interloquire anche con lui, pubblicando sulle pagine dello stesso quotidiano un mio intervento, dove ho fatto presente che le modifiche che avete apportato con questa finanziaria alla disciplina degli interessi passivi in materia di IRES penalizzano la grande platea delle piccole e medie società di capitali, a tutto vantaggio dell'*élite* delle grandi società e degli istituti di credito. Le piccole imprese, che costituiscono parte significativa del tessuto economico del Paese e di quella classe media che state cercando di mettere in ginocchio come se fosse un nemico da combattere, di fatto vengono utilizzate nell'ambito di questa manovra quale polmone finanziario per consentire l'incentivazione fiscale delle loro sorelle maggiori, evidentemente, a vostro giudizio, più meritevoli. Tale mia affermazione ha comportato nei giorni successivi, sulle pagine dello stesso giornale una piccata replica dello stesso dirigente, per spiegare che le mie tesi erano prive di giuridico fondamento. In realtà, per l'amministrazione finanziaria sarebbe stato meglio che questa replica non avesse avuto luogo e chi parla ha immediatamente respinto al mittente le incaute critiche che gli erano state rivolte! Nel formulare le mie considerazioni, mi baso infatti soltanto sulla rigorosa lettura dell'impianto normativo attualmente vigente e di quello prospettato da questo disegno di legge finanziaria. Con la finanziaria che stiamo esaminando viene, infatti, prevista l'abolizione di due meccanismi (la cosiddetta *pro-rata* patrimoniale e il cosiddetto *thin capitalization*) che oggi limitano la deducibilità degli interessi passivi, ma tali meccanismi si applicano, rispettivamente, soltanto alle società che possiedono partecipazioni e alle società con un fatturato superiore alla soglia prevista per l'applicazione degli studi di settore. Nessun effetto positivo consegue dunque per le tantissime società di capitali con un fatturato fino a 7,5 milioni di euro e che non hanno partecipazioni, in quanto non fanno finanza, bensì vera attività industriale e commerciale. Queste società, però, a fronte dell'eliminazione di meccanismi che già ora non le riguardano, vengono assoggettate al nuovo meccanismo di indeducibilità degli interessi passivi. Un meccanismo in base al quale gli interessi passivi (che le imprese sostengono per finanziare la propria attività, spesso per sopravvivere prima ancora che per crescere) risultano deducibili solo nel limite del 30 per cento del reddito operativo lordo prodotto. Se dunque io sono una società di capitali che fattura più di 7,5 milioni di euro, gestisce partecipazioni societarie di rilevante valore e consegue utili molto elevati, massimizzerò il beneficio fiscale rappresentato dall'eliminazione dei meccanismi che prima avrebbero potuto penalizzarmi e dall'introduzione di nuove limitazioni che comunque non mi toccano (perché grazie ai miei utili elevati, come ad esempio quelli delle banche e di alcune grandissime aziende italiane di questi ultimi anni, potrò comunque avere diritto alla deduzione di tutti o quasi i miei interessi passivi). Ecco che allora potrò davvero godermi in tutta piacevolezza la riduzione dell'aliquota IRES dal 33 al 27,5 per cento. Se invece io sono una società di capitali che non fattura più di 7,5 milioni di euro, che non fa finanza e che ha un'incidenza molto alta di indebitamento sul proprio reddito operativo lordo (sono certamente queste la maggior parte delle piccole imprese nazionali), scoprirò amaramente che anche con un'aliquota ridotta al 27,5 per cento pagherò più IRES di prima, in quanto su di me si applicheranno solo gli effetti negativi delle modifiche alla disciplina degli interessi passivi, e questi effetti negativi paradossalmente possono essere tanto più dirompenti quanto più la mia impresa è in difficoltà: poco reddito e tanti debiti. Dopo questa Dopo questa mia denuncia sulle pagine del più importante quotidiano economico nazionale, il Governo, nel corso del dibattito alla Camera dei deputati, ha attuato qualche leggero *maquillage* e sono state introdotte delle parziali attenuazioni del perverso meccanismo sopra descritto; ma l'effetto di travaso di fiscalità dal grande sul piccolo rimane, per le semplici quanto evidenti argomentazioni che sopra ho tentato di sintetizzare. Onorevole Sottosegretario, ho tentato nei pochi minuti a mia disposizione di aprire un dialogo con lei, sottoponendole problemi reali sui quali ora mi attendo una risposta vera; insieme a me la attende la miriade di piccole e medie imprese italiane che guardano con preoccupazione a questa manovra fiscale. Chi parla ha spiegato e documentato, credo in modo rigoroso, le proprie convinzioni. Vi sfido ora a dimostrare il contrario, ovviamente se ne siete capaci. *(Applausi

obiettivo. Credo che per quanto riguarda invece una serie di altre misure siano

ambientale e, nello specifico, le questioni che attengono all'applicazione del Protocollo di Kyoto e soprattutto ai piani di adattamento e di mitigazione per i cambiamenti climatici, dobbiamo dire con soddisfazione che linea che il Senato, in modo sistematico e sistemico, aveva indicato sia con il decreto collegato alla finanziaria sia appunto con la finanziaria stessa, è stata stata non solo riconfermata ma rafforzata, con l'introduzione di una serie di misure che riteniamo molto valide. Ciò riguarda specificamente il tema delle energie rinnovabili: vorrei ricordare che sono state

a decorrere dal 1° gennaio 2011, il divieto di distribuzione, di importazione e di vendita di tutte le lampadine ad incandescenza; lo stesso divieto per gli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica; le misure, di assoluto rilievo, in materia edilizia, che rappresentano a mio avviso un terreno di prova

certificazione che attesti il risparmio idrico. Sono elementi che ad alcuni possono sembrare di poco conto, ma che possono rappresentare davvero una svolta perché sappiamo tutti che l'Italia è, ahimè, indietro, e quindi in questi due anni stiamo facendo un lavoro di rimonta per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto, che è estremamente importante. Non basta però lo sforzo a livello è necessario che si proceda speditamente anche con la redazione dei piani energetici regionali da parte delle Regioni ed il contributo delle amministrazioni comunali è decisivo.

che hanno installato impianti fotovoltaici. Anche questa è una misura importante, che si accompagna alla

aumentare le speculazioni e le trasformazioni selvagge nelle nostre città. Noi invece dobbiamo procedere alla difesa dei nostri territori, al contenimento del consumo del suolo, perché anche questi c'entrano, eccome, con il Protocollo di Kyoto e i cambiamenti climatici.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, dedicherò questo mio intervento sulla legge finanziaria 2008 alle disposizioni riguardanti il settore energetico, uno degli snodi più caratteristici della manovra. Si tratta di un complesso di disposizioni distribuite in oltre 80 commi sui poco meno di 1.200 della legge, che delineano una radicale ristrutturazione della politica energetica del Governo, all'insegna di un marcato dirigismo, appropriato solo in economie di guerra. In seconda lettura, la Camera ha impresso a questa linea un grosso impulso, determinandone un cospicuo peggioramento. La filosofia generale sottesa a questa nuova politica energetica è ormai purtroppo quella totalmente prevalente in Europa, che attribuisce il progressivo riscaldamento del clima della Terra, osservato da qualche decennio, ad emissioni nell'atmosfera di gas serra dovuti ad attività umane, in particolare all'emissione di anidride carbonica per effetto della combustione di combustibili fossili, che prevede altresì a medio termine drammatiche conseguenze climatiche dovute a questo riscaldamento e che perciò considera perciò assolutamente necessari drastici e rapidi interventi di riduzione del consumo di questi combustibili fossili e la loro sostituzione con fonti rinnovabili;

parere) lo stato attuale delle conoscenze scientifiche sul clima e sulla sua dinamica, data l'enorme complessità delle interazioni energetiche fisiche e chimiche da cui è determinato, non consente né di attribuire con certezza la causa del riscaldamento climatico osservato all'anidride carbonica da combustione dei combustibili fossili (altre possibili cause o concause avanzate da autorevoli scienziati sono, ad esempio, una maggiore attività solare, in questo periodo ad un massimo storico, o l'influenza dell'agricoltura e della pastorizia che producono anch'esse importanti gas serra), né di prevedere quali saranno le conseguenze a medio e lungo termine del riscaldamento in atto. Al riguardo, la scienza non ritiene fondato il catastrofismo, sostenuto in Europa anche ad alto livello politico, secondo cui il riscaldamento globale in atto sarà presto accompagnato da gravi desertificazioni, imponente innalzamento del livello dei mari, rilevante aumento del numero e dell'intensità delle tempeste. La scienza, quella vera, rigetta queste affrettate attribuzioni di colpevolezza e queste false previsioni catastrofiche e rende perciò priva di fondamento e giustificazione la conseguente cura da cavallo che l'Unione Europea sta proponendo e che ora il Governo italiano sta applicando. La nuova politica energetica delineata da questa legge finanziaria è caratterizzata, innanzitutto, da una spropositata incentivazione della produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili. Le disposizioni principali sono quelle contenute nei commi da 143 a 157 dell'articolo 2. Le incentivazioni sono molto superiori a tutte le simili incentivazioni adottate negli altri Paesi europei. Un solo macroscopico esempio: per gli impianti eolici di taglia inferiore ai 200 kilowatt l'energia elettrica prodotta verrà pagata, nel caso dell'opzione in "conto energia", la bellezza di 30 centesimi di euro al kilowattora, cioè oltre quattro volte il prezzo dell'energia elettrica prodotta mediante combustibili fossili (7 centesimi di euro al kilowattora). Il Senato aveva approvato in prima lettura il valore già molto elevato di 22 centesimi di euro al kilowattora, ma evidentemente ciò non è bastato. Nella foga di legiferare, alla Camera si è stati qua e là sgangherati. Ad esempio, che vuol dire l'espressione «potenza nominale media annua» che ha sostituito l'espressione «potenza elettrica» votata al Senato? E che incentivazione avranno gli impianti eolici in "conto energia" di taglia compresa tra 200 kilowatt e la potenza nominale media annua di 1 megawatt (che verosimilmente sono la maggioranza)? Il costo di questa eccessiva incentivazione - che assommerà presto a svariati miliardi di euro l'anno - sarà pagato dalla platea degli utenti del sistema elettrico mediante prelievo automatico sulle bollette (con la voce A3), prelievo poi gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Si tratta a tutti gli effetti di un'imposizione assai simile a un'imposta fiscale, che ha però il pregio, agli occhi del Governo, di non aumentare il dato della pressione fiscale, così come oggi è calcolata dall'ISTAT, come ha gentilmente informato la settimana scorsa il sottosegretario Lettieri rispondendo qui al Senato ad una mia interrogazione. Ma gli utenti della bolletta elettrica dovranno anche pagare altri cospicui costi. In primo luogo, il costo di tutte le innovazioni sulla rete elettrica di distribuzione necessarie per consentire il pronto allaccio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, innovazioni rese obbligatorie dai commi 164, 165 e 166 dell'articolo 2. Si tratta di oneri tutt'altro che trascurabili, che tuttavia non risulteranno evidenti all'utente in quanto compresi nella fattura dei produttori di energia elettrica. In secondo luogo, per effetto della disposizione di cui al comma 146 dell'articolo 2, gli utenti del sistema elettrico dovranno pagare i costi dovuti al fatto che i produttori di energia elettrica sono tenuti a vendere un *mix* di energia elettrica di doppia provenienza, da combustibili fossili (o fonti energetiche ad essi per questo fine assimilate) e da fonti rinnovabili, con una quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinnovabili attualmente pari al 3,05 crescente annualmente, fino al 2012, dello 0,75 per cento: un incremento annuale enorme. Anche questi maggiori costi saranno nascosti nella fattura della fornitura di energia elettrica; nascosti, ma presenti. In sostanza, per effetto di tutte queste disposizioni il costo dell'energia elettrica è destinato ad aumentare in modo molto rilevante. Ciò avrà pesanti effetti depressivi sullo sviluppo del Paese, sia a causa della diminuzione della competitività del nostro sistema produttivo conseguente a questo scriteriato aumento di un fondamentale costo di produzione (già altissimo per l'Italia a causa della nefasta rinuncia all'energia nucleare), sia a causa della perdita di potere d'acquisto del cittadino utente domestico oberato, oltre che dalle tante imposte e tasse esplicite, anche da queste similtasse gravanti sul kilowattora. Esprimo poi una viva preoccupazione per alcune disposizioni che scardinano la tradizionale e collaudata distinzione di competenze

con una dotazione annua di 40 milioni di euro? Non è questo un compito specifico del Ministero dello sviluppo economico? Per quale motivo è stato affidato al Ministero dell'ambiente, con le disposizioni di cui al comma 176 dell'articolo 2, il Fondo per la piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile? Non sarebbe stata più propria la collocazione di tale Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico o presso il Ministero dell'università e della ricerca? Termino questo mio intervento esprimendo una viva contrarietà circa tre ulteriori disposizioni marcatamente dirigistiche contenute nella legge finanziaria. Con il comma 289 dell'articolo 1 si dispone che a partire dal 1° gennaio 2009 i regolamenti edilizi devono prevedere, per il rilascio del permesso di costruzione di edifìci di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una «produzione energetica» non inferiore Mi manca il tempo per commentare adeguatamente una disposizione di tale gravità, imposta d'acchito *erga omnes* prima di una qualunque congrua verifica della sua utilità, della sua praticabilità e dell'effettivo aggravio dei costi di costruzione da essa determinata. Con i commi 139 e 140 dell'articolo 2 si dispone che a partire dal 2009 le benzine e il gasolio per autotrazione posti in vendita sulla rete nazionale debbano contenere almeno il 3 per cento di biocarburanti. Ulteriori aumenti di questa percentuale potranno essere disposti con decreto interministeriale. Nessun rilievo hanno in questa disposizione le perplessità sorte recentemente, a riguardo dei biocarburanti, circa la effettiva compatibilità della produzione di agroenergie in parallelo alla tradizionale, prioritaria e fondamentale produzione agricola di derrate alimentari, nonché circa la asserita neutralità niente affatto esistente come tale - dei biocarburanti in ordine alla produzione di gas serra. Con il comma 163 dell'articolo 2 si vieta, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la distribuzione e la vendita in tutto il territorio nazionale delle lampadine ad incandescenza. Al riguardo, solo un rapido commento. A parte la singolarità dell'inserimento nella legge finanziaria di una norma che certamente non ha effetto sui saldi di finanza pubblica nell'anno 2008, va osservato che le lampadine di minor consumo alternative alle lampadine ad incandescenza hanno raggiunto prestazioni paragonabili alle lampadine ad incandescenza solo in una parte dell'enorme varietà di forme necessarie per le varie esigenze di illuminazione. Non appare quindi corretto introdurre una tale dirigistica esclusione generale. In conclusione, questa nuova politica energetica del Governo, caratterizzata da un'impostazione radicale fino al fondamentalismo, noncurante delle profonde ripercussioni negative che avrà sull'andamento generale dell'economia del Paese, appare il prezzo che le parti moderate della maggioranza hanno dovuto pagare alle parti estreme per mantenere in qualche modo unita al voto una maggioranza talmente diversificata da rischiare il collasso. Si manifesta anche in questo aspetto la grave crisi del nostro bipolarismo. *(Applausi dal

prendo la parola per fare il punto su una questione che ha molto appassionato quest'Assemblea: la lotta agli sprechi e ai costi impropri della politica. Questo è stato un elemento centrale dell'iniziativa politica di Sinistra Democratica e delle altre forze della sinistra. Abbiamo inteso soprattutto - voglio ricordarlo brevemente - mettere in campo una strategia che puntasse non soltanto, per così dire, a far volare un po' di stracci, ma guardasse ai rami alti. Che quindi non si limitasse a tagliare un po' di indennità ai consiglieri comunali, a chiudere qualche comunità montana e cose di questo genere. ragionevoli e opportune, ma certamente non tali da dare al Paese un segnale di particolare rilievo e peso.

La prima: ridurre i componenti del Governo. L'abbiamo fatto nel solo modo costituzionalmente corretto. Respingo la censura che sarebbe debole la scelta di applicare la nuova regola a partire dal prossimo Governo. Governo. Non si determina una crisi di Governo per legge, non si pone per legge un termine alla vita dell'Esecutivo. Ciò accade nel modo appropriato attraverso l'articolo 94 della Costituzione: questo l'ho già

per stabilire il precedente che al Parlamento è consentito decidere. Qualcuno sembrava dubitarne - ovviamente sbagliando - e il precedente potrà dunque tornare utile per il futuro. Infine, la terza: la questione dei maxiemolumenti pubblici, del *top management*, dei grandi dirigenti e così via. Perché siamo voluti intervenire sul punto? Voglio lasciare qualche considerazione nel resoconto di questa seduta perché nelle convulse giornate che hanno visto la formazione della finanziaria non c'è stato un momento di riflessione pacata che spiegasse per intero il senso dell'iniziativa. Parto da una considerazione: il governatore Draghi ricordava qualche tempo fa che il nostro Paese vede dei salari troppo bassi. Recenti studi dell'IRES CGIL dimostrano come il reddito reale dei lavoratori sia stato negli anni recenti pesantemente decurtato. In questa tendenza alla compressione del reddito da stipendio o salario troviamo pienamente gli apparati pubblici. Oggi il «posto pubblico» non consente più, come un tempo, una serena appartenenza a quella che avremmo definito la piccola o media borghesia. borghesia. Oggi il pubblico dipendente oscilla pericolosamente vicino alla soglia di povertà, soprattutto se monoreddito con famiglia. È un personaggio che entra in pieno nella sindrome della quarta settimana. È fra coloro che rischiano di perdere la casa perché aumenta il mutuo a tasso variabile di pochi euro al mese. È tra quelli che non riescono più a mandare i figli all'università. Parliamo quindi di insegnanti, poliziotti, impiegati comunali e tanti altri, sono caduti nelle classifiche del reddito e nella capacità di offrire ai propri figli un'adeguata occasione di mobilità sociale. Proprio di recente si ricordava su un grande giornale nazionale come questo sia stato storicamente nel Paese un elemento di forte coesione, che oggi sta venendo meno. Queste cose le sanno tutti. Quel che invece non tutti sanno è che nello stesso tempo in cui ciò accadeva, per una fascia non piccola di maxiburocrati e di dirigenti alti e altissimi, le retribuzioni sono schizzate verso l'alto, talvolta moltiplicandosi addirittura nell'arco di pochi anni. La proliferazione di enti, società a partecipazione pubblica, autorità, pseudo-autorità, mezze autorità di ogni tipo e caratura, ha ampliato in misura incontrollabile questo fenomeno, con passaggi addirittura eclatanti. Ne cito uno, non perché sia particolarmente censurabile, ma perché è veramente emblematico. Dalle relazioni della Corte dei conti risulta

il Paese che ha i salari più bassi d'Europa. Ma è anche il Paese con i privilegi più alti d'Europa. E'un Paese ad alta diseguaglianza. Vediamo come e perché è potuto Un tempo gli emolumenti pubblici trovavano un fondamento necessario nella legge. Tutto passava, prima o poi, in un modo o nell'altro, attraverso un confronto parlamentare. Tutto era visibile, pubblico, discusso e assoggettato ad un controllo sociale effettivo. Poi abbiamo privatizzato gli apparati pubblici. Ed è accaduto che per la generalità degli apparati pubblici, degli impiegati e dei funzionari, si è passati ad una contrattazione collettiva, da una parte pubblica e da una parte privata. La contrattazione collettiva ha sostanzialmente un grado di pubblicità e di visibilità non lontano da quello dato da un passaggio parlamentare. Ci sono confronti, scioperi, se ne discute, se ne scrive sui giornali. Si sa,

di cui nessuno sa nulla. Una trattativa sostanzialmente invisibile. Non sappiamo chi stende il contratto, chi ne definisce il contenuto, chi stabilisce le regole, i *benefit*, i vantaggi e gli svantaggi. E questa non è cosa da poco. Proprio la trattativa invisibile ha consentito l'esplosione di una fascia di megaretribuzioni pubbliche, di cui nessuno è stato fin qui veramente consapevole. E troviamo qui una vera e propria questione di *governance* di sistema. Come facciamo a sapere che in quella trattativa invisibile l'interesse pubblico, quello che ci riguarda tutti, sia davvero salvaguardato? E come si concilia il valore dell'imparzialità, del buon andamento, con la trattativa privata di emolumenti, *benefit* o quant'altro? Come definire il giusto e corretto rapporto tra politica amministrazione? Non potrà accadere per caso che questi valori diventino una moneta di scambio, una posta non dichiarata sul tavolo delle trattative ? E su quel tavolo dov'è la posta dell'autonomia e dell'indipendenza dei dirigenti? Non sarà messa in gioco perché in una piccola clausola scritta in basso a destra ci sono 50.000 o 100.000 euro in più? Si tratta di questioni che mettono

È per questo che abbiamo messo in campo l'allora articolo 91 del testo Senato, oggi comma 43 dell'articolo 3.

Ma potremmo ricordare al ministro Mastella che è stato fatto in molte occasioni. Il legislatore può certamente intervenire sui contratti in corso. Basti pensare alla legge sull'equo canone. Siamo intervenuti su milioni di contratti in corso e nessuno ha mai pensato che si applicasse solo alla scadenza di quelli in atto. Siamo intervenuti sulle assicurazioni,

manovra di finanza pubblica tesa a ridurre le spese. Abbiamo fatto delle eccezioni. Abbiamo, escluso, ad esempio le attività professionali. Voglio

un intervento scioccamente moralistico o pauperistico, ma abbiamo voluto porre una rilevantissima questione, che è un punto di *governance* di sistema.

pertanto, le ulteriori iniziative da assumere. Vorrei restasse a verbale in quest'Aula che consideriamo il ripristinato testo del Senato - l'ex articolo 91 ed oggi articolo 3,

stato fortemente modificato da quest'Assemblea in prima lettura rispetto all'iniziale stesura del Governo e - aggiungo - nel merito, a mio avviso, fortemente migliorato, oggi torna in questo ramo del Parlamento

per il 2009 e 270 per il 2010. Cioè, al di là del merito, si dimostra, insomma, che il Parlamento non si limita solo ad autorizzare nuove spese ma, il lavoro delle competenti Commissioni, reperisce nuove risorse; il che dimostra che, rispetto al binomio risanamento, equità e sviluppo, che è fondativo del programma del Governo Prodi, il rigore non è solo una prerogativa del Governo, come allo stesso modo, aggiungo, l'equità e lo sviluppo non dovrebbero essere solo l'esigenza di alcune parti politiche ma di tutto il Governo e di tutta la maggioranza. Noi rivendichiamo, ad esempio, alla sinistra, alla nostra parte politica, di aver puntato in questi mesi a misure di risarcimento sociale a favore dei più deboli, misure certo che hanno comportato un aumento di spesa, penso all'aumento delle pensioni minime, penso al programma per l'edilizia residenziale pubblica, penso al *bonus* per gli incapienti, alla lotta al precariato, che proprio con gli articoli definiti in quest'Aula è stata fortemente assunta come priorità, penso al tema del Fondo sociale o alle misure in favore dei giovani o dei ceti deboli in relazione all'affitto, come per alcuni versi alla stessa misura sull'ICI ad altre ancora. Noi facemmo bene, a mio avviso, a non accettare l'iniziale impostazione del ministro Padoa-Schioppa che prevedeva nuove uscite solo come prodotto dei tagli di spesa, ma invece di siamo posti il problema della crescita e il problema dell'aumento della domanda interna. Penso al tema del credito d'imposta per l'occupazione a tempo indeterminato nel Sud, un tema sul quale io vorrei richiamare l'attenzione del Governo, dato che è presente il sottosegretario Sartor che ha molto partecipato ai nostri lavori e che ringrazio: per anni il Mezzogiorno, che pure in questa finanziaria non è presente come sarebbe stato giusto, è stato oggetto, e dico volutamente oggetto, di politiche derogatorie, sia dal punto di vista attraverso lo strumento prevalente dell'accordo di programma, sia dal punto di vista addirittura salariale, e ricordo il tema dei contratti d'area. Ebbene, finalmente è finita una fase che, in nome di un'esigenza di lavoro, faceva diventare il Mezzogiorno terreno di scempi urbanistici (e qualche mostro ancora rovina le nostre coste e i nostri territori), o terreno di sperimentazione della reintroduzione del salario d'ingresso. Il Mezzogiorno è un'area, come il resto del Paese, dove bisogna creare occupazione stabile in settori produttivi e avanzati. Inoltre, a proposito Villone è stato molto efficace parlando dei costi della politica, a partire dalle norme per l'abolizione degli enti inutili, la limitazione delle consulenze, le assunzioni discrezionali ma soprattutto il tetto agli stipendi dei *supermanager*, dove si conferma, nella sostanza, la norma elaborata dalla Commissione bilancio del Senato e fortemente chiarita e richiamata nell'intervento del collega Villone. Queste misure, ecco la prima conclusione del mio ragionamento, sono di fatto le uniche che in questi anni hanno contribuito alla crescita con l'aumento della domanda interna, e hanno contribuito alla crescita, ovviamente, pur nei limiti che la crescita ha avuto e in qualche modo hanno limitato i danni rispetto all'aumento delle tariffe, delle tasse comunali e di tutte quelle situazioni che obiettivamente - basta sentire qualche inchiesta televisiva - fanno di questo Natale 2007 un Natale per molti settori delle nostre popolazioni più povero povero e più difficile rispetto a quello dell'anno precedente. Allora, altro che utilizzo dell'extragettito solo per ridurre il debito! Ma com'è possibile? Si voleva arrivare

bene, credo la maggioranza ma soprattutto noi che veniamo dal mondo del lavoro, il Paese, conosciamo quelli che non arrivano alla terza settimana, conosciamo quelli che per il precariato si dibattono tra assenza di futuro e povertà assoluta o relativa che sia. Sappiamo di tutti coloro che rischiano la vita ogni giorno per la mancata prevenzione contro gli omicidi sul lavoro. Ebbene, tutti questi soggetti, che pure non hanno ottenuto finora da questo Governo - del quale siamo parte

Ebbene, per tutti questi soggetti la finanziaria è certamente un primo passo - a mio avviso non del tutto sufficiente - verso l'equità e lo sviluppo:

- è stata sostanzialmente confermata alla Camera dei deputati. Di questo voglio ringraziare il relatore Legnini e tutti gli altri componenti della Commissione bilancio. Vorrei allora soffermarmi su tre punti che ritengo utili da segnalare. norma che introducemmo al Senato finalizzava le maggiori entrate tributarie alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare nel 2008 mediante l'incremento della misura della detrazione sul reddito da lavoro dipendente,

del 20 ottobre scorso, nella finanziaria vi è stata l'irruzione della questione salariale, come - per altri versi - della questione della precarietà. Oggi bisogna andare avanti

di lavoratori, dipendenti delle piccole imprese, nei settori dell'artigianato o in aree dove il sindacato è debole, a seguito di un simile meccanismo di abbandono della contrattazione nazionale, non si troverebbero più nelle condizioni di poter crescere in un Paese dove c'è una politica industriale.

- la percezione del dramma salariale è così forte, ma le politiche finora decise sono ancora troppo deboli e lavoreremo perché il tema del recupero salariale nel 2008 diventi realmente prioritario. Voglio brevemente soffermarmi inoltre sul tema delle politiche sociali. Anche qui, è inutile girarci intorno: il combinato congiunto dei tagli agli enti locali e l'aumento di alcune tassazioni locali ha determinato che quasi tutti i Comuni italiani, anche per via della riduzione del fondo nazionale per le politiche sociali operata dai Governi precedenti, hanno subito una contrazione dei servizi, soprattutto di quelli di prossimità: penso all'assistenza domiciliare agli anziani, al problema dei minori abbandonati e al grande tema dell'immigrazione e dell'accoglienza, segnalato, ad esempio, dal senatore Bonadonna con riferimento alle difficoltà di garantire diritti civili ad alcune popolazioni come quelle dei romeni. Ebbene, c'è una novità: mentre si raddoppiano i fondi per la non autosufficienza - ed è positivo

infatti ormai da anni che, per tutta una serie di motivi procedurali e passaggi in Conferenza Stato-città, prima della metà di maggio questi fondi non arrivano alle Regioni, le quali non le ripartiscono ai Comuni prima dei mesi di settembre-ottobre. Ma come si fa, in Comuni che hanno problemi finanziari enormi, soprattutto problemi di cassa, quando si tratta di portare avanti appalti triennali (penso ai settori dei minori o al settore dell'assistenza domiciliare agli anziani, penso all'assistenza all'*handicap* e alle case famiglia), a a mantenere gli impegni in primo luogo con i soggetti deboli, ma anche con le agenzie del terzo settore che erogano un servizio quando, per effetto di questa catena, non ci sono le risorse Si crea una situazione difficile che in molte città del Mezzogiorno (penso a Napoli), combinato con il problema del Patto di stabilità, ha determinato un disagio soprattutto ai più deboli, ma anche ai lavoratori di tali agenzie. Questa norma credo sia giusta! Infine, due ultime notazioni,

in Commissione bilancio al Senato della Repubblica. Credo che sia stato un bene e non certo perché qualcuno sul "Corriere della Sera" ne ha parlato, ma perché era evidente

il tema che si è posto è etico e morale nel nostro Paese. Se c'è un grande problema salariale, non possiamo assistere senza una strategia a situazioni - a partire ovviamente dai parlamentari - dove c'è un guadagno che toglie ogni rapporto fra qualità del lavoro e retribuzioni. Anche noi che siamo tra quelli più aperti e più impegnati sul fronte della lotta ai costi impropri della politica consideriamo un nostro successo aver evitato che si riducesse il numero dei

mai bisogna confondere la giusta lotta contro i costi impropri della politica con una sottovalutazione di quale risorsa sia per la democrazia il sistema della democrazia decentrata di base; un sistema che vogliamo difendere anche contro le tendenze a concentrare sugli esecutivi - siano essi sindaci, presidenti delle Province o le stesse giunte - tutti i poteri, esautorando i consigli comunali che invece sono l'espressione diretta dei cittadini. Ci dispiace però, in questo quadro, che alla quella sugli oneri di urbanizzazione (ha bene accennato su questo versante la senatrice De Petris). Pur comprendendo le difficoltà dei Comuni, ritenevamo sbagliato dare una risposta (volutamente faccio un bisticcio di parole) sbagliata ad un problema reale. Non si può risolvere il problema della dei trasferimenti ai Comuni permettendo di spendere del tutto per spesa corrente gli oneri di urbanizzazione. Lo scorso anno ci fu un'apertura di quest'Aula; quest'anno si era ridotto al 25 per

talvolta c'è un mancato coordinamento che attiene al tema della legge finanziaria, troppo pesante. Nel provvedimento Bersani-*ter* si discuteva del problema delle ferrovie e l'eventuale liberalizzazione di alcune tratte profittevoli; liberalizzazione di tratte profittevoli a cui Rifondazione Comunista e la Sinistra fortemente si oppongono, come si sono opposte alla privatizzazione della Tirrenia in nome di un principio della garanzia del trasporto pubblico e anche della copertura di tutte le aree del Paese, perché non v'è dubbio che liberalizzare il servizio ferroviario su tratte profittevoli, quelle che

a determinare un'indagine su questo aspetto. Per fortuna ieri sera in Commissione il Governo ha accolto un ordine del giorno del relatore Legnini, da me e da noi fortemente condiviso, che invita il Governo a non procedere ad alcuna opera di liberalizzazione nel settore fino all'approvazione da parte del Parlamento di una disciplina organica in materia e in particolare delle disposizioni per l'accrescimento dell'efficienza e della concorrenza, previste nel decreto Bersani. Queste sono, in sintesi estrema, alcune delle questioni che ci sembrava utile precisare e che sono i temi della verifica verifica chiesta, che non è, come talora in passato è stato, un problema di formule, di alchimie. Esistono, certo, problemi di riforma elettorale. Dal nostro punto di vista esiste il problema della rappresentanza democratica del Paese e dell'autonomia delle forze della sinistra rispetto ad un meccanismo che, più che privilegiare i programmi, rischia di privilegiare quello che in Aula qualcuno ha definito un bipolarismo coatto

a coloro che in questi anni hanno rischiato di perderla per la mancata presenza di una politica attiva sul lavoro e sul *welfare* e, soprattutto, rendere possibile, attraverso la verifica, magari con punti programmatici più limitati, di portare avanti un programma per la crescita e l'equità del Paese.

Qualcuno, del resto, l'ha definita quasi una finanziaria ottocentesca. A qualunque richiesta si è data risposta

In particolare, mi soffermerò sull'università e sulla ricerca scientifica; anche in questo caso non vi è un indirizzo nel merito. Si va avanti a forza di improvvisazioni (vedi il 10 per cento del Fondo per la ricerca scientifica cui illustri colleghi

No, perché i precari sono quei 200.000 della pubblica amministrazione, soprattutto quelli che ancora devono vincere il concorso (perché quelli che ne hanno vinto uno non saranno assunti nella pubblica amministrazione). Sono i tanti portaborse, che rientrano dalla finestra in questa finanziaria; quelli veramente sono precari e verranno assunti nei ruoli, alla faccia della ricerca scientifica e dei nostri tanti giovani che attendono

Qual è la possibilità per quel docente di assumere? Nessuna. Quindi, lo tiene lì come precario, lo fa lavorare dieci-dodici ore al giorno, in attesa che arrivi un evento. L'evento qual è? Un posto di dottorato con concorso, se non ci sono nepotismi diversi, un posto da assegnista, o, in attesa che il ministro Mussi lo emani, un concorso nazionale per ricercatori.

di questo mese, nella trasmissione «Che tempo che fa», dice che non è vero - ma forse non ha letto l'emendamento del taglio orizzontale, che ha colpito anche la ricerca scientifica - e si vanta di 500 milioni di di euro in tre anni, il che significa ogni anno 166 milioni. Togliamone 90, e ciò che rimane non servirà nemmeno a pagare gli aumenti di stipendio ai professori universitari. Altro che ricerca scientifica! Ma Prodi probabilmente non è al corrente di ciò e deve fare degli annunci. Però l'annuncio di Prodi a «Che tempo che

Ebbene, cosa pretendiamo da questo Paese? Il nostro è un Paese che sta rinunciando completamente ai suoi valori, non solo culturali, ma anche etici e morali. Del resto, il messaggio culturale è solo quello amplificato dai *media*, dove rubare, delinquere, uccidere, diventano meriti per poter fare carriera, diventare ricchi ed andare avanti nella vita. È questo il messaggio che vogliamo

significative modifiche nel campo dei trasporti, delle ferrovie, dell'autotrasporto. Ebbene, devo dire che in alcuni casi si tratta tratta di misure positive, in altri invece di misure che richiederanno correzioni ed anche qualche valutazione politica. Voglio partire subito dall'innovazione positiva contenuta nella norma sulla quale (voglio ricordarlo) anche qui al Senato, prima in Commissione bilancio e poi qui in Aula, avevamo richiesto una svolta

che dopo aver a lungo trattato e discusso con le città e le Regioni, nonché con le imprese di trasporto pubblico locale, ha finalmente avanzato una proposta stabile per dare sostegno e sviluppo a questo settore, di cui abbiamo fortemente bisogno per offrire ai cittadini un servizio migliore e nel contempo decongestionare le città dall'assedio del traffico motorizzato. Voglio ricordare che la misura che è arrivata al nostro esame in prima lettura conteneva già una quota significativa (500 milioni di euro) per il trasporto pubblico locale, ma il suo limite era proprio quello di essere destinata ad una sola annualità, quindi in futuro suscettibile di scelte diverse, e comunque oscillante sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

che devono effettuare le Regioni, un fondo stabile per lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Questo ammontare di risorse sarà pari a 1.748 milioni di euro nel triennio dal 2011 tale compartecipazione sarà definita con un decreto, entrando quindi a pieno regime. Si tratta di una misura positiva, che naturalmente non è esente da qualche rischio sull'efficienza della spesa, nel senso che

in un'efficienza dei costi per il servizio pubblico locale, in un effettivo sviluppo di offerta del servizio, nonché in un miglioramento della qualità e dell'innovazione dello naturalmente non avremmo ottenuto quello che con la norma ci ripromettiamo di fare. In questo senso, sono certa che la maggior parte delle Regioni vive e si impegna perché il trasporto pubblico locale vada in questa direzione. Questi sono anche gli impegni che le Regioni hanno assunto alla cabina di regia a Palazzo Chigi, ma credo che serva di più e che occorra un quadro di regole, regole, da discutere in Parlamento con il disegno di legge che il Consiglio dei ministri avrebbe già approvato, proposto dal Ministro dei trasporti, proprio per definire un percorso di efficientamento e sviluppo del servizio. Se dal lato delle risorse con questa misura tale percorso trova un'adeguata e stabile copertura, un punto di svolta per il nostro Paese e per le nostre città, al contempo occorre sia siano garanzie reciproche sulla qualità e l'efficienza di questa spesa, all'interno di un quadro di regole definito. Il secondo tema che vorrei affrontare, che è stato modificato nell'*iter* alla Camera, riguarda riguarda le ferrovie. Innanzitutto, desidero ricordare che all'articolo 2, comma 252, si destinano maggiori risorse (104 milioni di euro) al contratto di servizio per la media e lunga percorrenza.

positiva. Non positivo - lo voglio segnalare - è che anche con questa manovra restano irrisolti due temi che pure, anche nel passaggio al Senato, avevamo segnalato al Governo.

pendono annunci di tagli in assenza di compensazioni da parte del Governo nei confronti delle Ferrovie dello Stato che deve esercire questo servizio. conseguenza, se da un lato abbiamo risolto un problema, non abbiamo ancora risolto - e mi auguro che nei prossimi mesi ciò avvenga - il problema dello sviluppo del trasporto regionale

pendolari". Dopo aver investito sulle reti, mentre sono in corso gli investimenti sui nodi (che hanno ancora un certo ritardo), nonché la velocizzazione di alcune linee del Mezzogiorno,

di un confronto e di un'approvazione, preveda uno sviluppo di questo segmento intorno al 23 per cento. Tutte queste ipotesi di sviluppo, che naturalmente sarebbero molto positive perché abbiamo bisogno di dare alternative all'abuso dell'automobile per i cittadini e le imprese, non avranno in realtà riscontro, al di là di ciò che sta scritto nei piani, se non si avvierà il piano di acquisto dei mille treni per i pendolari. Avevamo segnalato al Senato questa grave carenza. Alla Camera sono state risolte alcune questioni legate alle ferrovie, ma quella riferita all'avvio di risorse per l'acquisto dei treni

Innanzitutto, non posso fare a meno di ricordare e anche di stigmatizzare questo modo di procedere, ricordando che una norma di analogo tema

sono stati presentati emendamenti, svolte riunioni anche con il Governo per segnalare la necessità di correggere quel testo e di integrarlo, proprio per garantire un processo di liberalizzazione regolata nel settore del trasporto ferroviario

ed aziendale straordinario, che dunque richiede una accurata valutazione rispetto alla quale si era sostanzialmente arrivati ad un buon risultato. Ecco invece che con il comma 253 dell'articolo 2 della finanziaria al nostro esame

correzioni in corso di valutazione. L'obiettivo, e lo dico anche a nome del mio Gruppo, non è quello di

Naturalmente, so bene che c'è una forte attenzione dei privati al trasporto ferroviario profittevole e di questo non solo non mi stupisco, ma comprendo anche le ragioni. Credo che di per sé sia positivo che investitori privati, che fino ad oggi hanno ritenuto il trasporto ferroviario un settore sostanzialmente da chiudere e per nulla significativo in termini di offerta di servizio ai cittadini e alle imprese, trovino nel 2007 di nuovo interessante reinvestirvi, ritenendo quindi meno interessante investire solo nell'autotrasporto e nello sviluppo del trasporto stradale. Se da un lato questo processo è positivo e va incoraggiato, dall'altro credo che chi regola la cosa pubblica debba individuare un sistema di liberalizzazioni in cui

Voglio ora fare una riflessione insieme a voi sul tema dell'autotrasporto. Il testo al nostro esame aggiunge 50 milioni di euro, che sono il risultato del blocco irresponsabile esercitato dal mondo dell'autotrasporto, che (come è noto)

la politica. Se da un lato ho censurato il metodo di lotta utilizzato, che ha paralizzato il Paese, voglio però ricordare che alcuni temi che vengono posti da quel mondo sono giusti. quel mondo sono giusti. Quando il Governo Berlusconi approvò la norma che liberalizzava completamente le tariffe ed anche il quadro di regole in cui esercire l'autotrasporto, l'opposizione

le tariffe dovevano avere una loro progressione, proprio in relazione al fatto che per la lunga distanza doveva essere viceversa incentivato il trasporto via mare e ferroviario: si trattava di adottare una certa coerenza di regole per non sfruttare sfruttare chi esercita il lavoro di autotrasportatore e, dall'altra parte, per definire una politica di trasporti coerente nel quadro degli incentivi. Peccato (voglio ricordarlo in quest'Aula) che tutti quegli emendamenti furono bocciati

ribadendo che alcune misure al nostro esame sono senz'altro positive. Su altre misure credo sarà opportuno chiedere nuovi e maggiori impegni al Governo, nonché un quadro

Signor Presidente, oltre al mio commento su questa manovra finanziaria, mi consenta di iniziare il mio intervento tentando di rispondere ad alcune giuste considerazioni che la senatrice Donati ha appena finito di svolgere. Mi riferisco in particolare all'ultima parte del suo intervento, a quando ha ricordato il processo di liberalizzazione dei trasporti posto in atto dal Governo Berlusconi con grande attenzione e tempestività, inserito in un processo di sviluppo della rete delle infrastrutture del nostro Paese, che è condizione fondamentale perché il processo di liberalizzazione dei trasporti possa avvenire. La senatrice Donati dovrebbe forse ricordare con la stessa puntualità anche il sapore e la capacità drammatica che hanno avuto le diverse manifestazioni che si sono svolte nel nostro Paese nel tentativo di bloccare alcune di queste grandi opere. Una per tutte: l'alta capacità ferroviaria, che ha un ritardo di circa 20 anni nel nostro Paese. (che pure la senatrice Donati considera giusta, perché ho colto bene il senso del suo intervento nel valorizzare comunque le tante buone ragioni degli autotrasportatori italiani) non può essere distinta dalla violenza e dalla

Non si può parlare di trasporti senza parlare delle infrastrutture, delle strade, della nostra capacità infrastrutturale. Ricordo che questo processo è fermo da qualche tempo, soprattutto da quando questo Governo di centro-sinistra governa maldestramente il Paese.

culturale, economico e finanche psicologico. Ma il Capodanno degli italiani sarà anche peggio del loro Natale perché dall'inizio dell'anno cominceranno a scontare tutti i pesi della manovra finanziaria che ci si appresta in questa ennesima lettura del Parlamento ad approvare, ovviamente con il nostro voto contrario. Quest'anno, con i vari passaggi che il provvedimento ha dovuto superare in Parlamento, i poveri cittadini sono stati ulteriormente salassati,

e voi non state proteggendo gli italiani e il loro potere di acquisto, già indebolito dallo svantaggioso cambio tra lira ed euro fatto da un Governo come il vostro, composto da tanti di voi. È sempre un Governo di centro-sinistra che frega gli italiani, soprattutto i più poveri. Come diceva qualcuno più autorevole di me - l'illustre senatore Agnelli -, solo un Governo di sinistra può far ingoiare certi rospi al popolo. E così è. poi il senatore Ciampi, ex Ministro della Repubblica e soprattutto ex Presidente della Repubblica, che come sempre vi soccorre quando vi mancano i voti. sapete infatti che non avete una maggioranza politica in questo ramo del Parlamento e che potete approvare queste brutte leggi solo grazie al sostegno dei senatori a vita,

vota una legge finanziaria di mirabolanti spese dopo che per anni ha sottratto dalle tasche degli italiani tutto quello che poteva. Un esempio su tutti: il cambio tra la lira e l'euro, che è solo colpa sua, la cui responsabilità Ricordatevi cosa diceva Ettore Petrolini: «Bisogna prendere il denaro dove si trova: presso i poveri. Hanno poco, ma sono in tanti»*.* Voi applicate alla lettera questo triste aforisma. Prendete i soldi guadagnati a fatica dai cittadini, sottraendoli con un'imposizione fiscale crescente. Non dimentichiamo che il peso delle tasse sul PIL, quel prodotto interno lordo che gli italiani contribuiscono a creare, è aumentato di due punti percentuali da quando siete al Governo. Altro che diminuire le tasse. L'impostazione culturale, economica, del *deficit spending* prosegue e peggiora una finanziaria che molti hanno definito inutile prima di me, ma che io definisco dannosa. Dannosa perché continua ad applicare una vecchia, ammuffita, logica che, ad esempio, tutto il comparto lavoro continua ostinatamente a tutelare solo perché è già tutelato, vuoi con aggiustamenti alle carriere, premi, prebende, riconoscimenti e quindi inevitabili aumenti che da quest'anno ingrosseranno in modo esponenziale la spesa pubblica. Perché un aumento di stipendio, un riconoscimento alle carriere di chi ha già un lavoro, di chi ha già una carriera, sapete meglio di me che nessuno mai lo potrà interrompere e quindi, negli anni, si continuerà ad alimentare la mirabolante spesa. Ma non dovevate essere voi a diminuire gli stipendi ai super *manager*? Non dovevate diminuire quella vergogna che porta gli amministratori di Alitalia, ad esempio, a guadagnare centinaia di migliaia di euro l'anno, invece di prendersi centinaia di migliaia di calci, come vorrebbero tanti italiani, visto come hanno ridotto la nostra compagnia di bandiera? Vogliamo parlare delle ferrovie? L'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, che prima la senatrice Donati citava con tanta puntualità e precisione negli aspetti politici, è il paradigma di quel sindacalismo che ha smesso da tanto tempo di difendere gli operai. Oggi difende solo sistemi di potere e qualche volta privilegi. Il caso dell'Eurostar Lecce- Roma parla da solo, non c'è bisogno di aggiungere altro. Allora, prendiamo atto che i meriti che i meriti che hanno avuto questi *manager* non ci sono; ci sono per certo i loro grossissimi e ricchissimi stipendi. E questo non lo trovate assolutamente contrario a quella richiesta, che sale dal Paese, di una flessibilità sempre più protetta per quei giovani che devono affrontare questi tempi durissimi? Il processo di *flexsecurity*, così come viene definito nelle più moderne politiche del lavoro, per voi non comincia mai. E i giovani non possono essere liquidati da Padoa-Schioppa come semplici bamboccioni, perché a me sembra che bamboccione sia lui, forse abituato a stipendi d'oro di quel *gotha* della finanza che viene qui a farci lezioni, passa dal Parlamento, non eletto da nessun popolo, nominato da qualche Presidente del Consiglio amico. Ci fa una lezione e poi non è nemmeno capace di far quadrare quattro conti, perché in questa finanziaria tutti i conti sono saltati. È il costo della politica vero, diceva prima qualcuno, di questa vostra cattiva politica che è costata solo in questi 15 giorni di passaggio alla Camera dei deputati 6 miliardi di euro in più. Forse qualcuno di noi non si rende conto di cosa siano 6 miliardi di euro in più. Tutto questo solo per sorreggere la vostra maggioranza che non si regge più in piedi nemmeno con lo sputo. Il senatore Vegas vi chiedeva prima se lo conoscete questo Paese. A me sembra che soprattutto non conosciate gli italiani, ma state tranquilli che loro vi hanno conosciuto. Questa finanziaria, la vostra finanziaria, è infarcita di favori e contentini. Vi state Vi state preparando a sostenere una difficile campagna elettorale, ma rassegnatevi: questa volta gli italiani non li fregherete più; questa volta gli italiani hanno davvero imparato a capire che solo un Governo di centro-sinistra può impoverire a tal punto gli italiani, così come avete fatto.

ci ha restituito una manovra tremendamente gonfiata, certo non arricchita, ma sovraccaricata di ulteriori problematiche. Se a quest'ora del pranzo - un momento inevitabilmente sonnecchioso - mi si consentisse un'allegoria, direi che

ceste di polli, a caschi di banane, a sacchi di patate, a pecore, a montoni e a tutto quello che è possibile caricare su questo *omnibus* e, per giunta, con un rimorchio targato Camera dei deputati su cui sono state caricate molte altre problematiche che qui non erano state prese in esame. Se si potesse sorridere su una malinconica allegoria come questa, sottolineerei in esame ha veramente il sapore di un'ultima spiaggia, «una finanziaria da ultimo autobus della notte», come se domani non vi fosse più nulla da fare o da intraprendere.

Questo sentimento forse non è estraneo a molti Ministri e sicuramente anche a molti deputati e senatori che sostengono la maggioranza. C'è quasi la sensazione che non vi possa essere un domani per questo Governo, visto che ha voluto fare tutto oggi in maniera farraginosa, disordinata e - come è stato sottolineato da molti colleghi - perfino disastrosa per gli effetti che produrrà sulla vita e in particolare sulle tasche dei cittadini italiani. Infatti, l'incedere di questo *omnibus* sferragliante, lungo strade polverose, di scarsissima trasparenza politica, pone un primo inquietante interrogativo che molti illustri colleghi della Commissione bilancio hanno già anticipato (come la senatrice Bonfrisco poco fa e il collega Vegas prima di lei): chi pagherà

spese. Qualcuno dovrà dire ai cittadini italiani che questa finanziaria contiene norme destinate a sconvolgere anche i loro sogni e, primo fra tutti, quello di avere una casa. Questo è un altro elemento davvero critico. La finanziaria in esame ha compreso una serie rilevante di materie con alto contenuto non solo tecnico ma anche politico e umano senza svolgere

capaci di assicurare una produzione di energia elettrica alternativa e rinnovabile non inferiore ad un kilowattora per ciascuna unità abitativa. di una piccola centrale elettrica non più indicata, però, come un'esortazione o un consiglio a guardare al futuro, alle fonti alternative e rinnovabili, ma piuttosto come obbligo e una condizione ineludibile per ottenere la licenza edilizia. Bisogna dire agli italiani che questa finanziaria contiene un vincolo del genere per quanti stanno facendo progetti per farsi una casa o accendendo mutui per pagarne le spese relative. Occorre

se si vuole davvero favorire anche la nascita di nuove imprese, come dice il testo del disegno di legge, nel rispetto delle competenze regionali. Se il Governo ha deciso veramente di prendere in mano le sorti del turismo, che sta soffrendo di molti problemi, lo faccia restituendo agli italiani

al lavoro compiuto dalla Camera dei deputati che ha posto rimedio ai pasticci combinati in quest'Aula da una maggioranza che non aveva capito bene il problema.

ma siamo consapevoli che non è in questo settore che si può trovare una risposta definitiva e importante all'allarme sugli sprechi della spesa pubblica. Vi saranno riduzioni nel numero delle comunità e nelle indennità riservate ai componenti e, soprattutto, nel numero dei Comuni montani: saranno indicati come tali solo quelli che veramente lo sono, ma non

Si voleva mettere in crisi il sistema di *governance* sostenuto dai piccoli Comuni e dalle comunità montane. Lo denuncia oggi, in un'intervista lucida e coraggiosa, il presidente dell'UNCEM, Enrico Borghi, su un quotidiano romano: si voleva consegnare tutto quello che oggi appartiene alla competenza, alla sensibilità e alla tradizione dei Comuni e delle comunità montane ad aziende municipalizzate gestite da Roma. Mi sembra

a coloro che sono nati, vivono o hanno deciso di continuare a vivere in montagna. È veramente il caso di ripetere un antico *slogan*: ministra Lanzillotta, giù le mani dalla montagna.

in questo campo una colonizzazione vorrebbe dire barattare tutto il patrimonio di esperienza, di umanità, di storia e di cultura di cui la montagna dispone - con quattro spiccioli rappresentati, nella controproposta della ministra Lanzillotta, da una serie - peraltro ridottissima - di infrastrutture per la produzione di energia elettrica. È persino offensivo poter immaginare di andare in montagna con una proposta del genere e affrontare seriamente la gente e tutti coloro che amministrano questa zona. Non ho consigli da impartire a nessuno, ma mi permetto di rivolgerne

Recuperi soprattutto la capacità di confrontarsi alla pari, scendendo dal piedistallo sul quale sembra essere salita (non si sa in base a quali valutazioni) e affrontando direttamente questi problemi con le persone e le comunità che li stanno fronteggiando e li subiscono da soli. Inoltre, potrebbe imparare molte cose - ne sono certo - in tema di gestione di quei territori, di trasparenza politica e amministrativa, ma credo anche di rispetto della dignità delle persone che hanno scelto di vivere - in molti casi di sopravvivere - in condizioni davvero difficili e delicate in zone in cui altri non avrebbero il coraggio di farlo. Solo perché sono decentrati, lontani e spesso isolati, non sono certamente cittadini di serie B e rifuggono da questo tentativo di colonizzazione ma, soprattutto, da qualsiasi ipotesi di tutela che possa provenire da Roma. Questo è un appello che rivolgo alla Ministra con delega alla montagna e, signor Presidente, affido anche a lei: è stata celebrata la settimana scorsa

dall'alto delle montagne le soluzioni da Roma, non si troveranno mai né l'ascolto, né la condivisione della gente. *(FI)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, cari colleghi (per quelli che siamo anch'io voglio accodarmi al coro dei colleghi della mia parte politica che sono intervenuti non già nel criticare il disegno di legge finanziaria, ma nell'esaminarlo - per quello che è stato possibile fare - e nel mettere in rilievo le grandi incongruenze, gli obiettivi falliti, il fallimento totale di tutta la manovra di quest'anno. Vorrei soffermarmi su alcuni dati semplicissimi. Signor rappresentante del Governo, signor Sottosegretario, con il disegno di legge finanziaria siamo partiti il 28 settembre con 97 articoli; al Senato abbiamo raggiunto i 151 articoli; alla Camera dei deputati fortunatamente si è scesi, siamo arrivati a tre articoli, ahimè! - tre articoli con 1.301 commi e con 324 pagine. Non ho fatto questa indagine, ma credo che sia la legge finanziaria più voluminosa, la seconda, come suggerisce il collega che più di me l'ha studiata. Credo che egli esprimerà, come relatore al disegno di legge di bilancio, il suo voto favorevole ma non il suo parere favorevole, non la convinzione di aver operato nel migliore dei modi. Siamo partiti da 10,7 miliardi della manovra; il Senato l'ha fatta lievitare al 13 per cento (per la verità, il Senato come istituzione, ma soltanto la maggioranza ha determinato questa lievitazione di prezzi); siamo arrivati alla Camera a 16,7 miliardi, cioè abbiamo raggiunto più del 50 per cento di aumento della manovra iniziale, con delle coperture anomale; le ha riferite il ministro Padoa-Schioppa in Aula

dato. Abbiamo bruciato i 6 miliardi che il Governo si vanta di aver recuperato con una maggiore politica fiscale, che ci ha portato ad un aumento del 40 per cento rispetto all'anno precedente, che rappresenta il 2 per cento del PIL e lo abbiamo bruciato con una serie di regali per conservare questa maggioranza, per regalare a destra e sinistra una serie di provvedimenti che non servono allo sviluppo. Il dato è che la spesa corrente è fuori controllo. Questo è il Governo del "tassa e spendi"; questo è il Governo della sinistra, che a noi preoccupa enormemente. Non ci preoccupa come impegnati nelle istituzioni, ma come cittadini e noi siamo gli interpreti della gente. È vero, questo Governo non ha la capacità di poter avere un colloquio con la gente. Se ha dei Ministri che camminano con cinque - cinque, caro senatore Villone - macchine di scorta, con 12 persone di scorta, che non hanno più il contatto con la gente, è chiaro che produrranno una serie di provvedimenti che non sono finalizzati a creare sviluppo per il Paese, ma soltanto un substrato che possa mantenerli in essere e quindi avviarsi a fare demagogia e occupazione non finalizzata allo sviluppo. Nuove tasse, nuove assunzioni all'interno del pubblico; si sta creando una bomba a orologeria per i prossimi Governi,

noi abbiamo cercato di apportare qualche miglioramento. Avevamo ottenuto che l'Assemblea votasse un emendamento sulla permanenza

Diliberto si preoccupò anche di redarguire Dini perché questo avrebbe portato un aumento di spesa e dimenticava che l'emendamento da noi proposto modificava una volontà da parte del Governo di spendere 14 milioni

si provvede a rimuovere un comandante generale della Guardia di finanza ed il TAR annulla il provvedimento come se nulla fosse accaduto.

voi ci avete rattristato; avete distrutto il nostro piacere di sorridere, di muoverci. Girate in questi giorni per le città: nemmeno la forza di mettere le luminarie hanno avuto gli imprenditori! È questo il dato, non già perché non vi sono soldi ma semplicemente perché non vi è più il desiderio

tra le modificazioni che la Camera ha introdotto alla legge finanziaria, e di cui ha dato stamattina conto il relatore Legnini, ce ne sono alcune che colgono di sorpresa anche la maggioranza e rispetto ad esse il giudizio che formulo è fortemente negativo. Parlerò quindi solo o principalmente di questi aspetti della legge finanziaria. All'articolo per finanziare il sistema alta velocità‑alta capacità, ricompreso nella rete di trasporto ferroviaria europea, viene utilizzata a questo scopo una quota del canone dell'infrastruttura ferroviaria. Che cosa significa?

vedrà aumentato tale canone (poiché la sua attuale commisurazione è appena necessaria per affrontare i costi di manutenzione della rete),

Dunque, Trenitalia, società di FS in passivo, dovrà, con i suoi mezzi, finanziare Rete ferroviaria italiana, la quale trasferirà la risorsa all'alta velocità e all'alta capacità.

è stata riproposta pari pari nella formulazione bocciata dal Senato. È, questo, un atto di arroganza, che non posso attribuire all'intera Camera, non è stata introdotta nella discussione in Commissione, né nella discussione in Aula, ma nel maxiemendamento. Dunque, siamo di fronte ad un atto di arroganza di origine ministeriale. Evidentemente, il Ministro in questione, il Ministro delle infrastrutture, vuole ottenere questo risultato a tutti i costi; non capisce però (e questo è il punto su cui mi voglio soffermare) che introdurre tale modalità realizza proprio quella situazione su cui recentemente il Ministro ha tuonato. Ricorderete che non più di quindici giorni fa, in un convegno a Napoli, se non ricordo male, il ministro Di Pietro ha aggredito l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato accusandolo di utilizzare le somme che vengono trasferite alle Ferrovie dello Stato per finalità di finanziamento di interventi infrastrutturali al fine di coprire i buchi del disavanzo di esercizio delle Ferrovie stesse. Di Pietro, dicendo questo, poi si contraddice quando ammette che Rete ferroviaria italiana debba finanziare con il proprio canone l'investimento sulle infrastrutture. Quindi, egli indirizza il canone di di Rete ferroviaria italiana a fini di investimento e contemporaneamente lo stesso Ministro deve poi riequilibrare i conti di Rete ferroviaria italiana con delle ricapitalizzazioni, quindi con dei trasferimenti ai fini di garantire l'equilibrio dell'esercizio. Per cui, il risultato finale qual è? Che si danno dei soldi per riequilibrare l'esercizio di Rete ferroviaria italiana, la quale li traduce in canoni che vengono trasferiti all'infrastruttura per realizzare la rete dell'alta velocità, esattamente quello di cui il Ministro accusava l'amministratore delegato Moretti. Bisogna tornare indietro da questa determinazione. Al comma 253 si introduce il principio della liberalizzazione delle tratte ferroviarie

nelle quali gli introiti da passeggeri e da merci riequilibrano i costi di esercizio (le cosiddette tratte remunerative) remunerative) imprese ferroviarie che abbiano la licenza di esercizio ferroviario (quindi, imprese pubbliche o private, italiane o straniere, purché abbiano questa licenza) possono mettere i loro mezzi, i loro treni, sulla rete ferroviaria chiedendo il diritto di passaggio (la cosiddetta traccia oraria)

e colui il quale lo detiene attualmente non può utilizzare tutti gli *slot* liberi perché altrimenti si determinerebbe una condizione di monopolio. Dunque, sulle tratte che si reggono senza il contributo pubblico intervengono soggetti diversi da Ferrovie dello Stato.

Parteciperà a gare di servizio pubblico sulla rete debole per le quali è prevista la compensazione dei costi da parte del bilancio dello Stato. Dunque, il bilancio dello Stato (che oggi non lo fa) compenserà i costi della rete debole. Contemporaneamente, quello che oggi viene fatto da Ferrovie dello Stato (la compensazione della rete debole con i ricavi sulla rete forte) verrà trasferito a soggetti terzi che attualmente non ci sono sul mercato e che potranno essere i francesi, i tedeschi oppure, come si sente dire, i nuovi vettori ferroviari di Della Valle e Montezemolo, anche se questo dovesse avvenire solo nel 2010. tratta di una soluzione assolutamente aberrante, contraria agli interessi del Paese e della finanza pubblica

se non ci fosse la fiducia, io questo articolo della legge finanziaria non lo voterei e credo che anche altri insieme a me non lo farebbero. Ci farà la fiducia, e ciò assolverà tutti da questo compito.*(Applausi

Signor Presidente, uno dei primi indici di decadimento mentale è la perdita della memoria. La differenza tra noi e i pesci rossi è che il pesce rosso dopo circa due secondi non ha più memoria di quello che è successo, che gli italiani e i padani un po' di memoria ce l'abbiano. Ebbene, ricordo qualche affermazione di una persona che ci tiene sempre su di morale, perché tutte le volte che lo vedo penso, signor Presidente, che non è vero che gli italiani sono tristi:

«Dobbiamo impegnare bene quanto recuperato dall'evasione fiscale e cominciare a restituirlo con la diminuzione delle imposte. Questo è il mio obiettivo futuro». E conclude ovviamente: «È un impegno

e i soldi arrivano dal controllo di questo popolo di evasori; un popolo di poeti e quant'altro, ma soprattutto di evasori.

«Mia madre di 77 anni percepisce 800 euro al mese di pensione. Questo mese si è vista consegnare 80 euro in meno». Andiamo avanti. Si trattava di un pericolosissimo evasore.

Ma dove sono andati a finire i nostri soldi? In qualche assunzione, forse 50.000 dipendenti pubblici in più. Noi non abbiamo niente contro i dipendenti pubblici; tuttavia, Presidente, vorremmo sapere chi è che paga

che colpivano la povera gente. Con la finanziaria abbiamo ripristinato quasi la tassa sul macinato; anzi, fin peggio,

Però neanche lui è riuscito a non far pagare i costi dei presentatori e delle ballerine, che prendono milioni e milioni di euro. A chi li facciamo pagare? Alla sciura Maria? Sì, alla sciura Maria, perché ricordo che il canone si paga soprattutto nel Nord del Paese. La città di Varese, più piccola di Napoli (non me ne vogliano gli amici napoletani, per i quali proviamo un grande affetto),

ma dico ai politici, a me stesso, a questo Governo: come facciamo a correre se ogni tre per due arriva un calcio negli stinchi? Allora è meglio sedersi, stare fermi, cercare l'evasione, non fare niente, cercare il modo di accodarsi insieme a tanti altri furbi al carrozzone pubblico, pensando e sperando che ci sia una parte del Paese, un determinato ceto sociale che continua a tirare la carretta italica, attendendo che nel cielo e nel firmamento possa arrivare lo stellone. non ha tutte queste opportunità, non ha tutte queste *chance*. C'è una parte del Paese che invecchia e una parte del Paese più giovane, che invece non riesce ad avere

Lasciamo perdere i Verdi, che vi fanno passare alcune cose, dopodiché appaiono norme a favore dei palazzinari, se ne aumentano le possibilità: diamo da credere qualcosa, complichiamo la vita agli italiani e poi lasciamo che i palazzinari... PRESIDENTE. La invito Non tra gli incubi, ma la religione cattolica ci invita alla santità.

il passaggio alla Camera ha riservato ulteriori amare sorprese per l'università e la ricerca italiane. Già questa finanziaria doveva scontare il taglio,

determinarne il funzionamento e non sono stati ancora banditi i concorsi per associato e per ordinario. Siamo quindi veramente ad un punto di non ritorno, con un'università abbandonata a se stessa, è paradossale come l'unica luce in questo contesto di assoluto grigiore sia quell'emendamento di Alleanza Nazionale approvato in Senato, fra l'altro contro la volontà del Governo e della maggioranza, che stanzia 120 milioni di euro in tre anni per le borse dei dottorandi di ricerca. È evidente che la colpa non è solo del